Grazie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

è noto da tempo, le reti transeuropee rappresentano un insieme di infrastrutture di trasporto integrate, fondamentali e strategiche previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare, soprattutto, la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione europea.

2050, che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'Unione europea, e una rete centrale, che sarà realizzata entro il 2030 ed è basata su un approccio di corridoi che dovranno includere almeno tre modalità differenti di trasporto attraverso almeno tre Stati membri e prevedere anche l'accesso ai porti marittimi. In tale contesto, la rete centrale è articolata in nove corridoi principali, quattro dei quali interessano appunto l'Italia. Uno è il corridoio Mediterraneo che attraversa il Nord Italia da Ovest a Est. A tal fine, il completamento delle infrastrutture di collegamento risulta certamente essenziale per ridurre il *deficit* infrastrutturale italiano, sostenere la competitività delle nostre imprese nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo. Il nuovo asse ferroviario tra Italia e Francia - e, più nello specifico, tra Torino e Lione - rientra, come sappiamo, all'interno del corridoio mediterraneo. Noi di Fratelli d'Italia, insieme alla stragrande maggioranza degli italiani, da sempre siamo promotori e anche sostenitori della TAV, i cui principali obiettivi sono di diverso tipo. Vi sono sicuramente obiettivi di tipo economico, per rendere più competitivo il treno per il trasporto di persone e merci; di carattere ambientale, per ridurre il numero di TIR sulle strade; di carattere sociale, per connettere meglio tra loro e valorizzare le diverse aree presenti all'interno del nostro Paese.

i dati più recenti dicono che ogni anno, tra Italia e Francia, passano circa 3 milioni di mezzi pesanti e, se le previsioni dell'Osservatorio sull'impatto della nuova linea fossero rispettate, dopo 8 anni dalla sua apertura, si assisterebbe a un trasferimento di 20 milioni di tonnellate da strada a rotaia e di 38 milioni dopo 30 anni; in quella data, se il flusso di merci tra Italia e Francia rimanesse stabile ai valori di oggi, vale a dire intorno ai 40 milioni di

formali, è ben noto che, essendo questo un trattato internazionale, l'adesione dell'Italia al progetto non può essere sicuramente cancellata o modificata con un tratto di penna. Ogni giorno di ritardo penalizza non sono le Regioni del Nord che vengono attraversate dalla linea, ma anche l'Italia intera. Non è nemmeno il caso di ricordare come siano in gioco penali a carico

i trattati possano essere modificati o addirittura sostituiti. Sicuramente l'Italia non ci fa una bella figura. Aggiungo che fonti nazionali e comunitarie hanno stimato in 3,4 miliardi di euro gli oneri a carico dell'Italia in caso di sospensione definitiva della TAV, considerando i costi legati alla rescissione dei contratti, agli appalti già avviati, al ripristino degli scavi; chiaramente, oltre a tutto questo, sarebbero a carico dell'Italia anche le penali, come ho prima detto. La mancata realizzazione imporrebbe, infatti, anche la messa in sicurezza degli oltre 26 chilometri già scavati e l'adeguamento del tracciato del Frejus. Non è nemmeno il caso di ricordare i posti di lavoro in ballo per quanto riguarda quest'opera e il rischio di creare ulteriore disoccupazione:

tagliata fuori dalle vie dello sviluppo europeo, a vantaggio di collegamenti a Nord delle Alpi. Analogamente non dimentichiamo che - come ho detto prima - i porti di Trieste e Genova rischierebbero di veder

Lo stesso dicasi anche per l'Interporto di Novara, un nodo cruciale per le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, che proprio lì vanno a incrociarsi.

non solo piemontesi, ma anche nazionali, e da numerosi amministratori locali che hanno manifestato, a più riprese, la volontà e il massimo sostegno alla realizzazione dell'opera: ciò avrebbe dovuto far riflettere il Governo e indurlo a confermare la TAV come

affinché possa tenersi, sussistendo i presupposti di legge, un *referendum* consultivo sulla realizzazione del progetto TAV Torino-Lione nella stessa data nelle Regioni interessate dalla tratta nazionale del corridoio Mediterraneo: parliamo del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

trovare una soluzione che sarebbe l'ennesima novità, ovvero una mini TAV di cui chiaramente nessuno sa nulla.

d'Italia farà tutto ciò che è possibile per dare continuità a un'opera che riteniamo fondamentale e strategica per il nostro Paese.

gli avvenimenti dei mesi passati hanno evidenziato in modo inequivocabile come il Governo non abbia una linea precisa e univoca sul progetto TAV, anzi di come ne abbia troppe. Ciò vuol dire non averne nessuna. La confusione regna sovrana tra i due partiti di Governo che, come in uno spietato gioco di forza, continuano a tenere il punto. Da una parte la Lega sembra spingere per il sì; dall'altra, vi è il no tassativo e categorico del MoVimento 5 Stelle. Il ministro Toninelli taccia l'opera come inutile e dannosa. Il *premier* Conte Conte sceglie di non scegliere e, in virtù del ruolo di garante, continua semplicemente a prendere atto della volontà dei suoi sostenitori politici, per di più su un tema tanto importante per ragioni economiche e di relazioni internazionali. Non credete che, arrivati a questo punto, gli italiani abbiano il diritto di sapere cosa pensate del TAV? Non credete sia necessario, opportuno opportuno e giusto che ci diciate nell'Aula del Parlamento, luogo principe del confronto istituzionale, cosa intendete fare della vicenda? Non credete sia giunto il momento di smettere di eludere le domande a cui non avete mai voluto o - a questo punto - saputo rispondere? Sono tanti gli interrogativi rimasti in sospeso. Quanto si spenderà se si porterà a compimento l'opera? Quanti sono i costi in caso di recesso? A quanto ammontano le penali in caso di non completamento? Avete ignorato le nostre domande e continuate a farlo in maniera irresponsabile. Oggi dovreste invece iniziare a dare risposte: lo dovete agli italiani e anche al ruolo che ricoprite. Le assunzioni di responsabilità sono passaggi della vita politica; non è rimandandole che si dura nel tempo, che si va lontano e si diventa credibili. È più semplice sostenere il Governo quando si devono distribuire zuccherini, ma è più complicato quando bisogna esercitare responsabilità politiche: vero, colleghi? La tattica è chiaramente quella di perdere tempo. Tuttavia, incombe a breve l'appuntamento dell'11 marzo, data entro la quale il consiglio deve sbloccare i bandi per 2,5 miliardi di euro per il *tunnel* di base, pena la perdita di 300 milioni di euro di finanziamenti europei. Anche se questi bandi possono essere revocati entro sei mesi - come ha seraficamente dichiarato il ministro Toninelli corre il concreto rischio di perdere finanziamenti europei, di dover restituire i fondi già concessi e di essere estromessi dalla ripartizione per i prossimi cinque anni: non è roba da poco. Perdere tempo, continuare nel gioco del rinvio, guardare solo ai singoli interessi elettorali è la sola strategia che sa usare il Governo, oltre a a quella delle chiusure. Chiudono grandi opere come la TAV o il Terzo valico, si chiudono i cantieri per sistemare strade, sottopassaggi, piste di aeroporto, ferrovie urbane, metropolitane e ponti, mentre un fantomatico decreto sblocca cantieri ha difficoltà a venire alla luce e stessa sorte tocca alla riforma del codice degli appalti. Tutto è bloccato. Crescono i timori e l'economia rallenta. Il Governo dispone sempre la chiusura, per non cominciare mai niente. Chiusure, contrasti, incertezze, rinvii, *referendum* della base e quant'altro sull'opera in questione: di fronte a questo stallo, la Commissione europea ha fatto sentire la propria voce, rimarcando il concetto che la linea Torino-Lione è un progetto importante non solo per la Francia e per l'Italia, ma per l'Europa nel suo complesso. Quella a cui assistiamo inermi è una crisi di credibilità, risultato inevitabile, dato dall'assenza di chiari e decisi provvedimenti di politica economica e industriale. È una crisi di credibilità certamente accentuata dalla posizione assunta nei riguardi della linea Torino-Lione. Non fare la TAV non vuol dire solo rinunciare a posti di lavoro e investimenti importanti, che possono rilanciare l'occupazione, lo sviluppo e il ma significa soprattutto condannare il nostro Paese a una sfiducia da parte del mondo delle imprese e a un ruolo marginale nei mercati internazionali. Un numero crescente di cittadini e imprese, lavoratori, associazioni, amministratori, sindaci, esponenti politici di tutta Italia chiedono, con sempre maggiore forza, il completamento della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. La verità, ormai innegabile, è che i reali ostacoli alla realizzazione dell'opera sono da imputare alla caduta verticale dei consensi del MoVimento 5 Stelle nei confronti dell'altro *partner* governativo, testimoniata dalle recenti elezioni regionali, oltre all'avvicinarsi delle elezioni europee e, soprattutto, all'impossibilità di mantenere fede a tutte le mirabolanti promesse fatte in campagna elettorale, che tolgono al Movimento qualsivoglia intenzione di fare ciò che si prospetta essere il meglio per il Paese e fare invece ciò che torna utile al Movimento Siamo passati da dichiarazioni che alludevano alla volontà di trovare soluzioni tecniche, con l'analisi costi-benefici, a frasi del tipo: «Troveremo un accordo politico»; il tutto senza rendersi conto che non solo si cadeva in contraddizione con quanto sempre sostenuto, ma che si conferma quanto sostenevamo da tempo e cioè che la soluzione alla questione TAV è tutta politica. politica. Altro che analisi costi-benefici: basta prendere in giro gli italiani! Mi chiedo se, qualora non ci fossero state mobilitazioni di piazza delle opposizioni e dei cittadini rispetto a questo vostro atteggiamento irresponsabile, la TAV sarebbe oggi un nodo politico da sciogliere. L'analisi costi-benefici sulla TAV Torino-Lione è stata oggetto di pesanti critiche per i gravi difetti logici

sociale attesi dalla realizzazione della stessa in termini di maggiore interconnessione del Paese con il sistema delle reti TEN-T europee, di incremento degli scambi commerciali e di maggiore mobilità per i cittadini. Lo stesso ordine degli ingegneri di Torino, riappropriandosi nel ruolo di tecnici che gli compete, parla nella sua controanalisi costi-benefici di errori e semplificazioni che hanno abbattuto i benefici e ingigantito i costi. Il tentativo è stato quello di dimostrare, al di fuori delle regole che disciplinano la redazione di una corretta analisi costi-benefici, che l'opera avrà un costo ampiamente superiore a quanto preventivato. Il documento non valuta invece se l'opera riesce a raggiungere lo scopo per cui è stata decisa e non calcola in modo analitico e completo i benefici monetari (ambiente, salute pubblica, sicurezza, mobilità) che sono a fondamento di qualsiasi investimento pubblico. Una seconda stesura dell'analisi richiesta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione delle critiche sollevate sul testo, ha ridotto l'impatto negativo dell'opera da 7,6 miliardi a 2,5 miliardi, confermando l'inadeguatezza e i difetti logici contenuti nel primo *dossier* costi-benefici. È chiaro dunque che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe sottoposto al Parlamento e al Paese, nonché al Governo francese e all'Unione europea, un'analisi costi-benefici palesemente infondata e oggetto di successivi aggiustamenti da parte del Presidente del Consiglio che, per uscire dalla situazione di evidente contrasto fra le forze politiche della maggioranza, ha recentemente espresso un parere positivo sull'ipotesi di realizzazione della cosiddetta mini TAV, appoggiando la proposta avanzata dalla Lega come progetto originario della TAV Torino-Lione. Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, la velocità della risposta economica e la competitività del nostro Paese dipendono in buona misura anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità di un Governo di guardare al futuro e dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto il resto dell'Europa e capace di creare crescita. I recenti dati diffusi dall'ISTAT sull'andamento della nostra economia rendono ancora più urgente l'avvio e il completamento di importanti investimenti pubblici. Colleghi, è un intervento in grado di incidere nei prossimi anni sulla crescita dei posti di lavoro, sul tasso di sviluppo del nostro Paese e non da meno sulla credibilità della nostra politica. Siete pagati per decidere: potete farlo e oggi fatelo.

dei poderi e, quindi, creare le condizioni perché il Corridoio Lisbona-Kiev potesse partire.

dall'Unione europea per una grande infrastrutturazione ferroviaria di tutto il sistema dell'Unione, con gli assi Est-Ovest e Nord-Sud. Ed è stata la scelta fatta dall'Italia di dare sviluppo, di creare opportunità per le nuove generazioni, per essere più ricchi e non più poveri. Questa è stata la scelta. TAV significa collegare Spagna, Francia e Italia fino a Kiev. 170 miliardi di interscambio con i Paesi Ovest, con la Francia e i Pirenei. TAV può significare, in futuro, andare fino a Pechino: non deve sfuggire che la Cina ha un grande piano di infrastrutturazione, che ragiona anche sulla Via della seta. Apprezzo il ragionamento, che ha fatto proprio ieri una parte del Governo in missione in Cina, di valutare attentamente e condividere il percorso della Via della seta,

La parte Torino-Lione della TAV è un piccolo pezzo in mezzo che serve a collegare e a essere centrali per stare meglio rispetto ad altri. Vorrei ricordare che, qualora ciò non avvenisse, il transito verrebbe spostato laddove c'è stata la discussione a fine anni Novanta e inizio anni Duemila, quando la Germania voleva il collegamento

Ed è stata una battaglia di questo Paese, dall'estrema destra all'estrema sinistra, unite, perché allora si capì che l'essere al centro e non alla periferia significava creare davvero le condizioni di sviluppo. Le economie tra Lione e Trieste, complessivamente, creano 1.200 miliardi di prodotto interno lordo: territorialmente, sono tra le più alte del mondo.

sta tra l'essere al centro o alla periferia. Sta nel fare degli altri porti, Genova e Trieste, l'attracco naturale dei traffici mediterranei e tra Est-Ovest. Altrimenti, solo con un Nord-Sud (anzi, con un Sud-Nord, in questo caso) avremmo traffici semidomestici per l'Europa. Vogliamo che l'Italia delle nuove generazioni non sia l'Italia dei pensionati o del reddito di cittadinanza, salvo che, senza giovani che pagano, si va verso il Venezuela. Questa è la realtà, se non ci sviluppiamo. Questo è il motivo che ha portato il Governo il Governo Berlusconi, nel 2004, a ratificare i primi accordi internazionali. Permettetemi anche, essendo piemontese, di fare un richiamo storico,

i nomi che hanno caratterizzato il *boom* produttivo e industriale del nostro Paese. Questo è il dato. Questo è il significato. Ma leggete anche la discussione del Parlamento di Roma, che è istruttiva, allorquando i contrari alla galleria del Gottardo sostenevano che non aveva senso che fosse pagata per il 70 per cento dall'Italia, dal momento che la galleria del Gottardo era tutta, al 100 per cento, in territorio svizzero. Anche questo è istruttivo.

Eppure, allora i nostri predecessori decisero di andare avanti: capirono che significava lavoro. Dal Nord Italia si fermò l'esodo verso gli altri Paesi (principalmente, a quei tempi, il Sud America).

e un ancor più complessa componente politica. Su questo tema non voglio essere ipocrita: è evidente che le due forze che governano il Paese partono da due posizioni diverse

Sta passando il messaggio di un Governo del no e di un bloccare le opere, dando la responsabilità prevalentemente a una componente della maggioranza,

a proteggere il nostro Paese e a prevenire credo che sia una cosa molto utile. Da questo punto di vista, il dibattito anche televisivo e mediatico che si sta facendo sul TAV certamente non ha paragoni rispetto a quello che avremmo dovuto fare su quel grande piano proteggi Italia *(Applausi dal Gruppo M5S)*su cui abbiamo investito tantissimi soldi. Non una volta ci è è stato chiesto di parlare di quell'elemento, mentre ogni giorno ci viene chiesto di parlare di un piccolo tratto di un corridoio transfrontaliero che già non arriva a Lisbona (dal momento che il Portogallo ne è uscito) e che già vede altri Paesi che stanno uscendo da questo progetto. Ciò non perché

penso ad esempio al fatto che la trazione stradale sta compiendo degli sviluppi molto più veloci rispetto a quella ferroviaria. Rispetto a questi temi, molti Paesi stanno facendo una riflessione

e di normativa, semplicemente utilizzando politiche logistiche, trasportistiche e di intermodalità che prima non si utilizzavano. È in questo modo che si produce lo scambio nodale, non facendo nuove infrastrutture. *(Applausi dal Gruppo

non hanno una visione negativa sull'opera, ma semplicemente hanno preso dei dati che sono quelli del 2011, perché è questo il modo corretto di rapportare le due nessuno è stato interrotto. Fate terminare.

nella letteratura scientifica delle scienze dei trasporti ci sono filoni accademici che ritengono lecito inserire pedaggi e accise nel calcolo, mentre altri ritengono che non vada fatto; questi elementi questi elementi erano previsti già all'interno delle analisi costi-benefici del 2011 dell'osservatorio. Da quel punto di vista, c'è coerenza totale tra l'analisi costi-benefici di allora e quella di oggi. Cambia che ci sono numerosi dati in più rispetto all'andamento dei trasporti e ovviamente il dato finale è stato modificato: l'analisi costi-benefici ci dice che quell'opera è profondamente in rosso, se vogliamo usare questa metafora.

All'interno di quel contratto di Governo abbiamo inserito semplicemente una cosa: una ridefinizione integrale dell'accordo Italia-Francia, una ridiscussione integrale del progetto. Rispetto anche all'interesse di entrambi i Paesi su quest'opera, ritengo che ci siano diverse perplessità. Anche la posizione della Francia non mi sembra che sia così chiara. Quindi andare a ridefinire con la Francia integralmente il progetto credo sia la cosa migliore che questo Governo possa fare.

credo che il dibattito di questa mattina dovrebbe cercare in qualche modo di fare lo sforzo di riportarci alla riflessione e al ragionamento su alcuni dati.

anche tutte le discussioni, i dibattiti, gli osservatori e gli aggiustamenti che ci sono stati negli anni hanno evidenziato sempre una serie di problemi di fondo. La questione fondamentale

cercato di portare acqua al suo mulino e ha trasformato questa discussione in una discussione ideologica. Voglio dire con estrema chiarezza qual è il punto di vista che noi cerchiamo di rappresentare in questo ordine del giorno.

hanno una ferrovia a binario unico, per cui tutti utilizzano ovviamente sull'autostrada e ne pagheremo i costi anche dal punto di vista sociale ed economico chissà per quanto tempo. Avrei quindi voluto veramente sognare e discutere in quest'Aula

dell'Atlantico già non c'è più dal punto di vista del Portogallo, per non parlare poi dell'arrivo a Kiev. Abbiamo visto in questi anni una riduzione drastica dei traffici su quell'asse.

portare ad aumentare la possibilità e la capacità della linea storica esistente. Tutto questo non è stato fatto, come non è stata affrontata un'altra delle questioni fondamentali che dovrebbe essere alla base della programmazione e della progettazione di qualsiasi opera, soprattutto sotto il profilo dei trasporti: sto parlando del Piano generale dei trasporti e della logistica.

Noi invece abbiamo iniziato una discussione molto accalorata in merito all'Alta velocità Torino-Lione insieme a quella sul Ponte sullo Stretto: vorrei ricordarlo a tutti, perché erano gli anni d'oro della legge obiettivo, di cui paghiamo ancora le conseguenze (perché siamo dovuti arrivare fino al 2016 per superarla, ad eccezione Quelli erano gli anni d'oro in cui bastava che si bucasse qualsiasi cosa: si potevano bucare le montagne, perché magari c'erano altri interessi, per cui si era inventata la legge obiettivo, con il *general contractor*, che ha creato molti problemi

seria su cosa avrebbe comportato fare investimenti infrastrutturali di ammodernamento in tutto il territorio italiano, soprattutto al Sud.

una crisi di 150.000 posti di lavoro. Forse non me ne ero accorta; probabilmente avevamo comandato. Invece non è così e lo sapete perfettamente. La crisi occupazionale che si è creata è avvenuta

produce in termini di posti di lavoro investire nelle piccole e nelle medie opere che riguardano davvero la comunità, invece di concentrarsi solo su una grande opera che ci fa discutere molto e che probabilmente corrisponde

che mi è concesso non mi consente di approfondire, quindi dirò in modo chiaro che è noto che nel nostro Gruppo vi sono posizioni diverse: per quello che mi riguarda, dico subito con chiarezza che sono per la realizzazione dell'alta velocità. Lo dico senza infingimenti e vorrei motivarlo con tre brevissime argomentazioni. C'è intanto la necessità di confermare gli accordi internazionali e, da questo punto di vista, c'è un problema di credibilità. la via scelta dal contratto di fare un'analisi costi-benefici evidentemente con molta chiarezza non ha funzionato e non funziona. Io trovo che la discussione che stiamo facendo ora, in questo momento, sia un po' kafkiana. Ieri sera c'è stato un vertice che non ha concluso niente; concluso niente; bisognerebbe capire qual è in realtà la direzione di marcia.

ci fossero un quadro di priorità e una strategia sul tema della programmazione trasportistica e logistica; ma non c'è niente di tutto questo. Tutta la discussione ormai si riduce a come si gestisce il tema del consenso in relazione alle elezioni europee. Questo è un danno per il Paese, anche prescindendo dai diversi punti di vista in relazione a quest'opera. Infine, visto che il tempo mi incalza, rimane sempre e comunque un grande tema: come l'Italia incrocia i grandi corridoi europei. Da questo punto di vista, la figura che sta facendo l'Italia mi preoccupa.

che è in grandissima emergenza, e non può essere messo in contrapposizione con le opere indispensabili di ammodernamento.

ma di tutto questo non vi è traccia, nemmeno nel dibattito tra le forze politiche di maggioranza, tantomeno è data a quest'Aula la possibilità di discutere. Questa è la mia posizione, che mi sembrava giusto e corretto evidenziare.

come ricordava il collega Errani, discutiamo di una questione sulla quale il Governo non ha fatto ancora conoscere la sua opinione finale.

per bloccare l'opera è necessario abrogare due leggi, la n. 71 del 2014 e la n. 1 del 2017. Fino a che non si toccano queste leggi, il blocco dell'opera La seconda questione riguarda le verifiche costi e benefici che si sostiene - lo ha fatto per ultimo il capogruppo Patuanelli - essere state fatte soltanto di recente. È completamente falso: la prima risale al 2003 e la fece l'Unione europea, anzi la fece la BEI (una valutazione finanziaria sull'*incipit* delle opere) e la seconda al 2008 e ne fu protagonista il vice ministro Castelli, leghista, nel Governo Berlusconi-*quater*.

ad aderire al progetto imperiale cinese della via della seta. Benissimo: se partecipiamo ad un progetto di questa natura senza definire qual è la nostra strategia della politica estera e commerciale e, soprattutto, della rete logistica con cui l'Italia si presenta, noi rischiamo di aderire ad un megaprogetto perdendo completamente la nostra autonomia.

logistico per l'Italia. La domanda finale, allora, è qual è la strategia che il Governo italiano intende mettere in campo per essere competitivo e stare nel cuore dell'Europa, soprattutto mantenendo le proprie responsabilità sulle reti europee, che ci hanno visto firmatari e sottoscrittori con Governi di natura e caratteristiche completamente differenti.

*(PD)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, vorrei cominciare a sgombrare il campo da alcune questioni sull'argomento di cui stiamo ragionando. Il problema di cui parliamo non è andare da Torino a Lione, argomento sollevato da alcuni detrattori di parte per minimizzare l'opera. Non è un problema locale, anche se poi lo diventa in un secondo momento e spiegherò alla fine dell'intervento il perché. La questione è, prima di tutto, nazionale e poi europea.

europeo. Se cancelliamo il corridoio, non finisce lì. Se non si costruisce la linea TAV tra Torino e Lione, si fa l'interesse della Germania con la Budapest-Lione

In secondo luogo, non solo favoriamo un altro Stato come la Germania, ma danneggiamo il nostro Paese facendogli perdere più di 800 milioni di euro di finanziamenti europei, di cui 300 milioni subito e facendo scadere i bandi TELT. Questi argomenti sono già stati affrontati

ciò è funzionale al ragionamento che sto sviluppando. Concordo con Salvini anche quando spiega che le infrastrutture servono per la crescita e che il TAV è più sicuro, più veloce, costa meno e inquina meno (ma anche su questo arriverò dopo), argomentando in linea con il mio pensiero.

e poi non è detto che sia a loro così chiaro il valore dello zero in rapporto alla virgola, visto che nella manovra della legge di bilancio nel rapporto *deficit*-PIL si è passati dal 2,4 al 2,04 con una *nonchalance* che faceva rabbrividire, pensando forse che gli italiani fossero un po' sciocchini e non cogliessero questo gioco delle tre carte. In terzo luogo, dire no al TAV significa - è stato ricordato anche adesso - non solo dover cambiare due leggi italiane, ma anche violare due regolamenti e comporta, soprattutto, la disdetta unilaterale da parte dell'Italia di un trattato, cosa per cui non esistono precedenti. Il tema della credibilità è serio in Europa perché la credibilità porta poi il rispetto.

perché in casi diversi noi siamo riusciti, grazie alla credibilità conquistata da ministri come Padoan, a farci rispettare. Credibilità, serietà,

Se queste cose sono ben chiare, lo dobbiamo allora dire. Lo dobbiamo dire con la stessa chiarezza con cui il ministro Tria, in una trasmissione televisiva qualche giorno fa, ha ammesso chiaramente - sono le sue parole - che nessuno verrà mai ad investire in Italia se il Paese mostra che con un cambio di Governo non si sta più ai patti: si cambiano i contratti, si cambiano le leggi e le si rendono retroattive. Lo ha detto il Ministro dell'economia, a lui ispiriamoci.

In un'epoca in cui è necessario evitare sprechi del denaro del contribuente, stabilire come allocarlo è sicuramente fondamentale. Lasciamo da parte le dure critiche al rapporto del gruppo di lavoro guidato dal professor Ponti, che in questi giorni hanno riempito i giornali e le trasmissioni televisive, anche se, dal mio punto di vista, una commissione come quella, senza doversi ergere a giudice imparziale, forse non dovrebbe nemmeno comportarsi come un avvocato, che deve dimostrare le tesi del cliente.

si dice - ai francesi, prima che la vedessero il Parlamento e una parte stessa del Governo, parla di un impatto negativo di 6.995 milioni di euro. La seconda, richiesta dal presidente Conte, ha ridotto l'impatto negativo a 2.225 milioni. Già la differenza è notevole, ma

c'è una domanda fondamentale sul trattamento di tasse e pedaggi. Viene infatti evidenziato come la diminuzione degli introiti per lo Stato nasca dalla diminuzione delle accise relative al transito su gomma e alla diminuzione delle entrate A questo punto mi pongo una domanda di altro tipo: è positivo o no lo spostamento da gomma a ferro? È evidente che questa è una domanda di carattere politico. C'è, però, un altro elemento ancora più strano. I No TAV sostengono sempre che si spendano tantissimi soldi per un'opera che verrà utilizzata da pochi. La relazione, invece, dice che quanto più l'opera attira traffico, se si considerano le conseguenze, tanto più essa è uno spreco. C'è, quindi, una contraddizione veramente pazzesca; infatti, portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, persino se ce la regalassero lo Stato ci perderebbe, partendo da quanto contenuto in quell'analisi.

risposta. L'analisi è stata costruita a livello europeo, ma si riverbera negativamente sul piano italiano. Soprattutto, gli stessi autori dell'analisi

Torino possa essere un punto in alto della cartina d'Italia. Mentre una volta lo sviluppo italiano era basato sulla logica del triangolo industriale Genova-Milano-Torino, recenti studi

che il problema non sono nemmeno più i numeri, non è la risibile analisi costi-benefici; il problema è l'idea di futuro che noi abbiamo. Un futuro che assomiglia pericolosamente al trapassato prossimo; magari fosse il passato remoto, quello citato da Pichetto

debbano pensare alle generazioni future *in primis*; non devono essere nemmeno sondaggisti con la necessità di uscire dalla contingenza, con la volontà di guardare quello che i cittadini vogliono in quel momento: devono tornare ad avere *vision*. Penso che il MoVimento 5 Stelle e la Lega abbiano

messa nel contenitore del contratto di Governo. La marmellata ha cominciato a fermentare. Volete un consiglio? Aprite il barattolo prima che i gas della fermentazione lo facciano scoppiare. Pensate al futuro del Paese invece che alle elezioni europee: non ve lo chiede il PD, non ve lo chiedono soltanto le piazze, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle attività produttive, Grazie

è veramente surreale, quasi ridicola, perché ad un'analisi costi-benefici puoi far dire esattamente quello che vuoi. Tanto è vero che ce ne sono due e ciascuna delle due dice una cosa contraria all'altra e, secondo me, ciascuna delle due afferma cose giuste e sbagliate contemporaneamente. Pensiamo, ad esempio, alle considerazioni sulle esternalità legate alla CO2. Non esiste un'informazione sul prezzo della CO2; varia da 30 a 120 sterline a tonnellata, secondo una stima del 2010 della Corte dei conti inglese, fino alle stime attuali della Commissione europea, unite sui cambiamenti climatici che afferma che tanto più il *budget* di carbonio scende, tanto più il prezzo della CO2 schizza a più infinito. Ciò è ragionevole. Il *budget* di carbonio è quello da considerare quando si decide di investirne una parte per realizzare qualcosa che ha un progetto di decarbonizzazione. Affidarsi a questi numeri, partoriti da analisi che, per loro stessa natura, non sono esatte, è una follia. Persino le scienze esatte non fanno questo. Per citare un signor nessuno, persino Albert Einstein ha prima supposto che la forza di gravità fosse un sottoprodotto della curvatura dello spazio-tempo e dopo ha cercato le conferme numeriche, non il contrario. Questo aspetto va tenuto in considerazione. Inoltre l'analisi costi-benefici è basata su analisi di mercato. Le proiezioni del libero mercato sui flussi di merci; dove sta la politica? Non è né dietro l'analisi costi-benefici, né dietro i parametri di tale analisi. In un'analisi

l'analisi costi-benefici ha dato un esito negativo in termini economici. Benvenuti. Guardate che è così sempre. Credete che il progetto AlpTransit, con i quattro *tunnel* (Lötschberg, Zimmerberg, Ceneri e Gottardo), abbia dato un'analisi costi-benefici positiva?

alla domanda sul perché la linea storica della Val di Susa è sottoutilizzata. Essa è sottoutilizzata perché il mercato ha stabilito che farvi passare delle merci su rotaia non è conveniente. Lo credo: il massimo carico è di 1.500 tonnellate in tripla trazione

il fondo. Esiste almeno un tipo di carro merci per trasporto motrici che non ci passa, per una questione di interbinario. È lo stesso motivo per cui chi prende l'alta velocità tra Milano e Roma a un certo punto si trova su un treno che va a 250 chilometri all'ora, perché l'interbinario scende da 4,40 metri (fino

i presidenti dei consigli di amministrazione delle ditte, che agiranno secondo il mercato. Nella seduta di ieri, il collega Bagnai ha giustamente detto che il mercato non è il perequatore di ultima istanza, ma è una variabile, che deve venire dopo scelte che dobbiamo fare a livello politico. Questa è la cosa su cui ragionare e pertanto questo tipo di opera deve essere inquadrato in una progettualità, come ha detto giustamente la collega intervenuta in precedenza. Al di là della mia posizione sull'opzione zero, vi invito a riflettere su questi parametri di base, perché la politica deve arrivare prima e non dopo.

e pertanto, ogni volta che cambia il Governo, come nei Paesi peggiori del Sud America, si rimettono in discussione le scelte fatte e approvate con Trattati internazionali. Questo è il dramma che sta vivendo l'Italia.

e noi vogliamo denunciarlo oggi. Questo immobilismo blocca l'Italia. A me dispiace citare il presidente della commissione tecnica, il professor Ponti, ma come si fa a dare credibilità a un professore che ieri ci ha comunicato che nell'analisi costi-benefici non vengono incluse le penali che si devono pagare nel caso in cui non si realizzasse l'opera? Siamo di fronte a un'analisi farlocca *(Applausi dal il professor Ponti non ha inserito nell'analisi. Cari colleghi, voi pensate che con questi stratagemmi e con queste scorciatoie potrete risalire la china? Io penso che dobbiate avere il coraggio di proporre un'operazione verità al Paese,

oggi state vivendo questo dramma: siete alienati dalla vostra assenza di identità, non sapete più chi siete. Siete al Governo o all'opposizione? Avete aperto alla società civile candidando nei collegi maggioritari tanti esponenti provenienti dalle professioni e oggi pagate questo scotto perché non avete maturato una cultura di Governo. Negli anni Sessanta la Democrazia Cristiana dovette lottare con un grande partito, il Partito Comunista Italiano, per la costruzione dell'autostrada del sole. Gli argomenti adottati in quegli anni sono gli stessi addotti dagli amici 5 Stelle: è un'opera pubblica inutile, che determina sperpero di denaro e poi la corruzione, questa maledetta piaga. Non è che si frena la corruzione controllandola, ma si elimina l'opera pubblica perché si ha paura. In quegli anni quelli erano gli argomenti, ma poi il Partito Comunista Italiano ha fatto un percorso, è maturato un convincimento nel governare il Paese, si è assunto quella responsabilità, ha avuto la metamorfosi, ma certo non è durata tre anni. Questo è ciò che paghiamo oggi, cari colleghi: un Movimento in profonda metamorfosi, che purtroppo fa pagare a noi italiani

perché era sperpero di denaro pubblico. Chi oggi avrebbe il coraggio di dire che nella Capitale d'Italia quell'opera sia stata un grande spreco di fondi pubblici? È questo approccio culturale, è questo approccio di Governo che a voi manca e che io auspico voi possiate maturare in questi anni.

dal Gruppo FI-BP)*. Non ne ha azzeccata una. Non ha fatto partire una sola opera. L'unica cosa che ricorderemo del ministro Toninelli (le *gaffe* le evito) è il pugno alzato al cielo in quest'Aula. Non ho altre immagini, non ho provvedimenti. Troppa fuffa

farci capire qual è la loro strategia nell'ambito del consesso internazionale. chiederete alla Francia un supporto e un sostegno nella elaborazione dei progetti. Non so quale sia lo stratagemma, ma vi dico, con estrema sincerità e schiettezza, che qualunque stratagemma voi oggi andiate a individuare questo non vi porterà a crescere nel consenso del Paese. Toglietevelo dalla testa. Non siete più credibili come forza di Governo. Dovete, necessariamente, fare un'analisi retrospettiva e introspettiva per capire chi siete. Quando la farete, forse tornerete ad essere credibili. Voglio capire meglio. Oggi voi chiedete alla Francia di aiutarvi e di aiutarci. Prima, però, andate in Francia, a Parigi. Parte la carovana del *leader* politico Di Maio insieme a Di Battista, che oggi è sparito. Prendete l'aeroplano, andate a Parigi, legittimate i *gilet* gialli, poi tornate e dopo ventiquattro ore subito smentite quell'operazione e oggi chiedete alla Francia di aiutarci. Ma con quale faccia? Con quale faccia?

Signor Presidente, oggi voteremo l'ennesima mozione in cui si cercherà di esaltare il temporeggiare. Altro che Quinto Fabio Massimo: voi ormai siete maestri. L'avvertenza che vi diamo è che, purtroppo, tutti i dati reali sono negativi.

Con questa modalità, il Paese non troverà mai alcuna forma di crescita e di occupazione. Con questa modalità, saranno purtroppo i dati reali che suggelleranno il fallimento delle vostre azioni politiche, perché, purtroppo, non siete credibili. *(Applausi Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il MoVimento 5 Stelle ha sempre manifestato, qui e altrove, la propria contrarietà alla realizzazione della linea ad Alta velocità Torino-Lione. Ci hanno sempre accusato di avere una posizione ideologica e infondata, ma l'analisi costi benefici ha dimostrato chiaramente a tutti che la nostra posizione era, ed è, fondata su solide basi e sulla conoscenza dei dati. Non si può dire certo altrettanto dei sostenitori del sì, che da anni accampano giustificazioni fasulle, fantasmagorici aumenti di traffico fino ad ora mai visti. Addirittura, si parla di saturazione della linea storica, che in realtà è utilizzata ben al di sotto delle sue possibilità, mentre la saturazione doveva essere il prerequisito per l'opera in base al primo accordo con la Francia. La posizione più ricorrente è anche la più interessante politicamente: dobbiamo andare avanti per non perdere i finanziamenti europei e far lavorare le imprese (sostenuto anche ieri dal neo segretario del Partito Democratico, Zingaretti, a Torino). Quindi, l'opera va fatta, non perché serve, ma perché ci danno una parte dei soldi per farla. Quindi, per avere qualche milione dall'Unione europea (comunque soldi pubblici, che in parte diamo noi all'Europa), ne spendiamo miliardi di nostri: e poco importa se serve o no. Vi sembra l'atteggiamento giusto e responsabile di chi in passato ha governato un Paese? Le risorse pubbliche vanno spese nell'interesse dei cittadini (e l'analisi costi-benefici dice che l'interesse pubblico non c'è) e non per fornire facili guadagni alle imprese che vorrebbero realizzare l'opera. Di infrastrutture necessarie, in Piemonte e nel resto di Italia, ce ne sono centinaia da finanziare e tutte più utili di un nuovo *tunnel*, dove c'è già una linea ferroviaria a cui servono pochi interventi migliorativi per renderla più competitiva. Una linea che, già oggi, può sopportare un aumento di oltre il 100 per cento del volume di merci trasportate.

contro i 60.000 che percorrono la tangenziale di Torino. Sono quelli i mezzi che dobbiamo togliere dalle strade. Quelli che percorrono le distanze medio-brevi e inquinano tutta la Pianura Padana. Consiglio ai colleghi che sono intervenuti prima di verificare meglio i dati prima di citarli a caso. Tutte le previsione di aumento del traffico merci sono disattese su tutto l'arco alpino. Si registrano la metà delle merci rispetto alle previsioni su cui era stata fondata l'opera trent'anni fa

Raccontano che senza questa linea saremmo tagliati fuori dall'Europa e che comprometteremmo il corridoio Mediterraneo previsto dall'Unione europea la tratta Lisbona-Kiev, che non esiste più perché il Portogallo si è sfilato già nel 2012 e senza pagare alcuna penale. Nulla di più falso, comunque, perché il corridoio Mediterraneo è costituito, per la maggior parte, da linee ferroviarie tradizionali e autostrade e non da linee ad alta velocità. Ne fanno già parte sia l'autostrada del Frejus che la storica linea ferroviaria Torino-Lione. Quindi, non tagliamo alcun collegamento internazionale se fermiamo la linea TAV e non lasciamo alcun buco nel corridoio Mediterraneo. Se non credete a me, potete verificarlo da soli, andando sulla sezione mobilità e trasporti del sito della Commissione europea, dove sono riportate tutte le tratte. Ma non possiamo certo infrangere l'accordo con la Francia, dobbiamo essere dei *partner* credibili. Solo che la Francia ha già spostato i lavori della sua tratta nazionale a dopo il 2038, ritenendoli investimenti non prioritari. E sapete perché il *tunnel* di base non l'ha invece ancora rinviato?

quella la rimandano al 2038. Non è strategica e la loro Corte dei conti dichiara la spesa non prioritaria per gli interessi del Paese. E non finisce ancora qui, perché questa fantastica opera ha un altro altro piccolissimo problema che la rende anche poco conveniente dal punto di vista ambientale. Sì, perché la temperatura nel *tunnel* di base si aggirerebbe intorno ai 50 gradi centigradi. Capite bene che non sarebbe percorribile dai treni e, quindi, andrà anche refrigerato. Pertanto, si vorrebbero costruire i due *tunnel* - uno per ciascun senso di marcia - come due enormi frigoriferi sotto la montagna, lunghi ciascuno

tema, ma non per importanza. Sapete oggi quanti treni merci viaggiano sui circa 1.000 chilometri di linee ad alta velocità già esistenti in Italia?

lo fanno sui convogli dello stesso tipo di quelli dei passeggeri (mi riferisco al treno ETR.500, ossia il modello precedente al Frecciarossa 1000). Quindi, se pensate che sia vero che sulla nuova linea viaggeranno *container* o i TIR direttamente caricati sui treni, vi sbagliate di grosso, oppure credete alle favole che ci raccontano da M5S)*. I colleghi di Fratelli d'Italia nella loro mozione scrivono che «il completamento delle infrastrutture di collegamento risulta essenziale per ridurre il *deficit* infrastrutturale italiano, sostenere la competitività delle imprese italiane e favorire una maggiore integrazione tra Nord e Sud del Paese, nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo; oggi la priorità a livello europeo è quella di garantire la continuità dei corridoi». Noi concordiamo, solo che il *deficit* infrastrutturale sta altrove: nelle linee mancanti per arrivare a Matera da Roma, o nelle linee a binario unico della Puglia o dello stesso Piemonte. E non c'è un collegamento mancante tra Torino e Lione, mentre tanti colli di bottiglia sul resto delle ferrovie italiane ci sono, eccome. Investiamo in quelli, allora, perché attraverso la linea esistente passano già sagome maggiori rispetto a quelle che poi possono attraversare il Piemonte e proseguire verso Genova. Ci sembra che, più che la nostra, la vera posizione ideologica sia quella di chi vuole il *tunnel* ad ogni costo, di chi usa questo argomento in maniera strumentale come arma di distrazione di massa per distogliere l'attenzione dai provvedimenti del Governo che stanno cambiando il nostro Paese:

lasciamo lavorare il presidente Conte, che è in riunione con i due Vice Presidenti del Consiglio e con il ministro Toninelli, e che intendono valutare in modo corretto l'analisi costi-benefici per trarne le conclusioni più giuste. Insieme troveranno la migliore soluzione, che sarà certamente quella che consentirà di tutelare l'interesse nazionale.

senatore Romeo, prevede la ridiscussione integrale del progetto, auspico anche a livello personale che, una volta conclusa questa discussione (cosa che spero avverrà molto presto), si andrà proprio nella direzione auspicata dalla senatrice De Petris. Ciò

Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, sono più di vent'anni che discutiamo della tratta Torino-Lione, ogni volta snocciolando dati, finanziando analisi sui costi, alcune utili e altre un un po' strumentali. Quello che è certo, però, è che nessuno in coscienza può dire di sapere oggi con certezza quali saranno le tecnologie, la società, il

il periodo di vita di un'opera come questa. Non lo sappiamo noi esattamente come non lo sapeva chi, a metà dell'Ottocento, realizzò il *tunnel* del Frejus. Nessuno allora poteva neanche immaginare quale sarebbe stata la tecnologia di oggi, lo sviluppo dell'elettronica, la capacità e la volontà delle persone e delle imprese di spostarsi, l'attuale livello del commercio. Voi che siete più giovani, se per caso vi incuriosisce, andate a vedere il dibattito e le polemiche degli anni Sessanta sull'Autostrada del Sole: si diceva che era un'opera inutile, che non c'era un livello di trasporti tale per costruire un'autostrada del genere. Oggi, francamente, credo che nessuno abbia dubbi sulla lungimiranza di quella scelta. Per questo la decisione è innanzitutto politica, una decisione peraltro già assunta. Ci troviamo a ridiscutere per l'ennesima volta con il 10 per cento dell'opera già realizzata. È un'assurdità per chiunque abbia un minimo di raziocinio. Le linee di trasporto sono state sempre, nella storia dell'umanità, corridoi di sviluppo economico e di comunicazione tra i popoli. Dovremmo smetterla di parlare della Torino-Lione: qui stiamo parlando perlomeno

non ha più nulla a che vedere con i fatti, i dati e le scelte. In questo senso, diceva qualcuno tanto tempo fa che prima di fare l'Appia nessuno viaggiava sull'Appia, giustamente; fatta l'Appia si è viaggiato sull'Appia. Questo è quello che vi dovete ricordare. Stiamo pensando a un'opera proiettandola a trenta, cinquant'anni, non è un'opera che guarda il presente, e anzi anzi si spera che la crescita economica, diversamente da quello che sta succedendo, aumenti la mobilità, i commerci, gli spostamenti e dunque dobbiamo farci trovare pronti.

il voto contrario su tutte le mozioni e ovviamente il voto favorevole sull'ordine del giorno presentato. Il Sottosegretario auspica che si vada poi nella direzione indicata dal mio ordine del giorno, ma nel frattempo la mozione di maggioranza ancora una volta cerca di non decidere e di prendere tempo.

a tutti che non si può pensare o illudersi di riuscire a tirare a campare, facendo partire le gare per poi magari revocarle,

per questo Paese.

Grazie

ambientalmente dannosi, gran parte dei quali va a foraggiare il trasporto su gomma e l'autotrasporto, quindi esattamente il contrario di quello che oggi i fautori del TAV vorrebbero venire qui a raccontarci.

visto che non è riuscita a convincere neanche il senatore Errani, che pure fa parte della sua componente nello stesso Gruppo, a sua volta Misto. È una tesi ardita, ma apprezzo

la realtà e la verità che possiamo trovare non solo dal presente, ma anche dalla storia. Negli ultimi cinque minuti, mentre ascoltavo i colleghi, ho guardato alcune date. È venuto fuori che nel 1839 - pensate - per la prima volta in Italia si costruiva una ferrovia, lunga solo pochi chilometri (7,25 chilometri).

che per fortuna erano state inventate, perché prima gli uomini andavano solo a cavallo. Ma si poteva forse andare solo a cavallo e non inventare neanche le carrozze. Poi un certo Benz,

E, se avessimo dovuto immaginare il costo delle strade per far camminare le vetture con quel motore a scoppio, perché non camminare sempre a piedi o con i cavalli? Ce n'era bisogno? Toninelli avrebbe avrebbe deciso sicuramente che il motore a scoppio era qualcosa che faceva male all'umanità e avrebbe continuato a dire che era meglio andare con le carrozze. i fratelli Wright nel 1903 decisero addirittura che si poteva volare e per la prima volta misero in cielo una macchina che veniva sollevata dall'aria e che, con una persona a bordo, faceva un piccolo tratto.

Ma perché non limitarsi ai viottoli di campagna? Costi e benefici? Non mi dilungherò troppo su quanto gli altri colleghi hanno detto e diranno, sul percorso incredibile dell'analisi costi-benefici, che prima era di 7,6 miliardi e che improvvisamente diventa di soli 2,2 miliardi al massimo di *deficit* e di impatto negativo. Non mi dilungherò nell'illustrare il danno enorme che il blocco degli appalti, cioè il blocco del TAV, provocherebbe. Dico che, oltre alle cose che hanno detto tutti (il ripristino delle aree, le penali, le mancate contribuzioni dell'Europa), io non credo sempre a ciò che

mondo opposte. Il resto sono chiacchiere. Ma plasticamente i cittadini hanno fatto vedere come la pensano. Da un lato, a Torino, ci sono state due grandi manifestazioni civili e pacifiche, per uno sviluppo controllato, certo, attento ai costi e attento acché nessuno rubi. Ma non è che per non far rubare non si fanno le cose. Dall'altro lato, le aree della sinistra più antagonista hanno dato vita in questi anni con violenza estrema al movimento No TAV, troppo a lungo accarezzato

anche se poi i voti li prendete per il reddito di cittadinanza che con i No TAV non ha molto a che vedere, considerato che molti sono figli di papà che non hanno bisogno di un reddito di cittadinanza. Mi meraviglio, però, degli amici della Lega. Voi sapete che noi abbiamo fatto e stiamo facendo un'opposizione patriottica. Vi abbiamo sostenuto nella politica sull'immigrazione, nonostante, anziché lavorare per il blocco navale che vi abbiamo ripetutamente chiesto di ottenere, vi siate fermati al no agli sbarchi, forse per non contrastare gli amici dei 5 Stelle. Così, di fronte al movimento

di fermare la legge sulla legittima difesa, voi tentenniate e consideriate possibile diminuire quello che i vostri elettori - i nostri comuni elettori - vi hanno chiesto? Possibile che, siccome a loro non piace la *flat tax*,

si possa ottenere con il No TAV e, dall'altro, quelli che credono invece che non si ferma il progresso, ma lo si controlla, lo si gestisce, lo si governa con onestà, con serenità, ma anche con scelte chiare, non con scelte mini. Infine, come se tutto ciò non bastasse, c'è un dato

se ha ragione chi la pensa come voi o come noi. Concludo, signor Presidente, dicendo che c'è una ragione che per me vale più di tutte le altre, il valore della parola data: dal Gruppo FdI)*. Chi mai investirà in Italia, se si potrà pensare che la nostra parola non vale niente, quando Toninelli decide che va cambiata?

Il forse esiste ancora nell'esito del vertice di ieri, che non ha deciso nulla, ed esiste ancora più chiaramente nella mozione presentata dai colleghi della maggioranza, persino a prima firma del presidente Romeo, che impegna il Governo a ridiscutere tutto. Siamo ancora al forse. È il caso di dire che - anch'io faccio una citazione latina - *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*. Mentre si entra in recessione tecnica, il mondo delle imprese di costruzione è fortemente in crisi. Due delle prime tre per fatturato rischiano di scomparire in questi giorni. Mentre tutto questo accade e gli organismi autonomi e indipendenti ci mostrano che le previsioni sul prodotto interno lordo vanno assolutamente riviste in diminuzione, qui si discute e ci si consiglia. Abbiamo visto una cosa imbarazzante: il sottosegretario Dell'Orco ha detto

- che, quindi, sarete costretti a rivedere. Vedremo in che modo e con quali strumenti. Servirebbe a questo punto un grande piano di investimenti pubblici. Lo sanno anche gli studenti di economia che a questo stato di cose bisogna rispondere in quel modo e, invece, si bloccano anche le opere già finanziate - vedremo anche come - che potrebbero dare sviluppo, aiuto alla ripresa del PIL e lavoro alle imprese. Ci vorrebbe un Governo illuminato che sappia programmare e decidere soprattutto; abbiamo, invece, un Governo tanto confuso che il ministro Toninelli non sa bene dove sedersi e si è seduto giustamente nei banchi del Senato, quasi che

perché ogni giorno che passa è un danno in più per il Paese. Questa Assemblea saprà avere un sussulto di autonomia e di dignità quando ne discuteremo e noi lavoreremo perché ciò accada. Il modo in cui il *dossier* sulla è stato portato avanti fin qui è l'emblema di una strategia fallimentare di questo Governo. È una strategia senza un punto di vista che guardi lontano e senza la capacità di affrontare neanche le cose dell'oggi, visto che domani bisogna decidere di far partire i bandi, se non si vogliono perdere 300 milioni di euro. Avete iniziato spacciando l'analisi costi-benefici, che era diventato una sorta di mantra, come una specie di strumento innovativo, dimentichi che solo su quest'opera se ne sono fatte una decina. A un certo punto avete detto di aver fermato i bandi, ma per fortuna non l'avevate fatto. È stato detto che non esiste l'inizio dell'opera. Mi è già capitato di dire

analisi costi-benefici, scelta con elementi così oggettivi che tutti coloro i quali ne hanno fatto parte, ad eccezione di un componente, si erano già dichiarati contrari all'opera. È come se, in un processo penale, la corte giudicante fosse costituita dai pm e non da persone terze rispetto allo stesso giudizio. È come se al liceo ci dessero un compito con la traccia chiusa: Dimostri il candidato che l'opera non è conveniente. Hanno lavorato come se direbbe Totò - a prescindere quest'opera non si dovesse fare. Questo è il modo in cui ha lavorato questa commissione, compiendo degli errori sui quali non voglio annoiarvi. Mi fermo proprio a quelli più evidenti. Si assume per assioma che l'infrastruttura costerà più del preventivato; si trascura la circostanza che di quel costo ben il 40 per cento è a carico dell'Unione europea. Si considera un costo per la collettività il minor utilizzo del carburante e dunque la riduzione delle accise: una follia. Quel che noi abbiamo detto essere un problema per l'ambiente e per l'inquinamento diventa, in questa analisi costi-benefici, un costo. Addirittura si considerano un costo i soldi in meno che le concessionarie guadagneranno attraverso i pedaggi;

di analizzare un'opera ferroviaria guardando ai danni che ne avrebbe, per conseguenza, un'opera stradale? si fosse deciso di non fare l'alta velocità in tutta Italia per i problemi che ciò ha determinato ad Alitalia: una vera follia dal punto di vista dell'analisi costi-benefici. di fronte ad un'analisi fatta dal punto di vista monetario e finanziario, che esclude completamente la valutazione dei benefici veri, quelli ambientali, in termini di salute pubblica, di sicurezza, di mobilità. Errori così marchiani che, dopo pochi giorni, su *input*, pare, di Conte, si è dovuto dire che c'era bisogno di una seconda stesura e sono stati richiamati in fretta e furia. Insomma, un'analisi costi-benefici più frutto di *fake news* e di analisi pregiudiziale, che non di studio serio, approfondito e scientifico. Concludo, Presidente, perché non voglio soffermarmi di più su un tema che pure mi appassiona. In economia, come è stato già detto, l'affidabilità è un bene primario. Non si investe in Paesi che non rispettano i patti, non si investe in Paesi in cui i Governi cambiano opinione

Gruppo PD)*. Per inciso, mi rivolgo al senatore Malan, che l'altro giorno ha fatto alcune affermazioni, molte delle quali condivisibili. Il PD e i nostri Governi sono sempre stati coerenti sull'opera; sempre, dal 2003 ad oggi, non c'è stato un momento in cui i nostri Governi abbiano avuto incertezze. Concludo davvero, Presidente. Seneca, nelle «Lettere a Lucilio», scrive che gran parte del progresso è nella volontà di progredire. Se questa volontà non l'avete, colleghi della maggioranza, fatevi da parte, mettetevi di lato, fermatevi: è l'unica cosa che possiate fare per il bene del Paese.

Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, come noto la Lega e il MoVimento 5 Stelle non si sono presentati alle elezioni del 4 marzo 2018 in coalizione e con un programma unitario. Per questa ragione, per dare stabilità al Paese e consentire il superamento dello stallo, è stato concordato e sottoscritto un contratto di Governo, allo scopo di disciplinare e indirizzare la futura attività di Governo. Tra i temi discussi, sicuramente le grandi opere hanno avuto il rilievo che meritano e, nello specifico caso del treno ad alta velocità Torino-Lione, su cui la Lega ha più volte espresso una posizione favorevole, si è ritenuto di dover procedere a un approfondimento. Obiettivo condiviso da entrambe le forze politiche è stato quello di rivedere il progetto e verificare la possibilità di realizzarlo risparmiando risorse e riducendo l'impatto ambientale. Ipotizzando un risparmio di un milione di euro, infatti, si libererebbero risorse da destinare ad altre opere prioritarie, consentendo così di risolvere problematiche presenti in altri territori. Daremo pertanto seguito, come prevede la mozione unitaria che abbiamo sottoscritto, a quanto previsto nel contratto di Governo, che ci impegna a valutare quest'opera, nel rispetto degli accordi internazionali. il traffico merci attraverso i valichi alpini italiani

che hanno detto che invece improvvisamente, da quando si era deciso di fare la linea ferroviaria, gli scambi e i traffici di merci erano in costante discesa. È qualcosa che sentiamo ancora oggi.

dicendo senza compromessi che ero, così come Forza Italia è sempre stata, a favore del TAV.

cioè diventati gli esperti del Governo.

Il fatto di considerare un costo aggiuntivo la diminuzione del traffico autostradale e, di conseguenza, gli introiti dei gestori delle autostrade e le minori tasse che lo Stato incassa, è veramente demenziale.

è veramente un altro elemento straordinario. Un altro fatto straordinario è che dell'analisi costi-benefici abbiamo sentito parlare fin dal primo giorno di insediamento del Governo Conte, il primo giugno 2018. Passati otto mesi, finalmente arriva l'analisi costi-benefici. Credo che ci potrebbero essere dei tempi minori perché se solo per fare l'analisi ci vogliono otto mesi,

Se non si realizzerà questa tratta, i grandi traffici di passeggeri, commerciali e turistici

Colleghi della maggioranza, le decisioni che prendete in questa sede le prendete voi e non i capi dei vostri partiti: siete voi che votate. Le decisioni che prendete qui non hanno effetto soltanto sui sondaggi o sui *like* di Facebook, ma hanno effetto sulla vita dei cittadini, per decenni. Per decenni, se si dice no a quest'opera, l'Italia sarà più povera e ci saranno meno

quando abbiamo votato la ratifica degli accordi con la Francia nel 2017, i tempi degli interventi sono stati contingentati incostituzionalmente: giusto per chiarirlo a chi si lamentava che si parlasse poco di questa opera in Aula. Bene, parliamone. Questa storia del TAV è intrisa di anomalie gravissime, di regole calpestate, a cominciare dalla repressione violenta attuata dai Governi precedenti a danno dei cittadini e delle cittadine della Valsusa. C'è C'è da domandarsi, infatti, come mai un popolo si compatti in questo modo, trasversalmente, dai giovani agli anziani, dal vigile al sindaco, contro un'opera che voi definite fondamentale, e che per vent'anni non si arrende, ma continua a lottare. Avete mai ascoltato le loro ragioni? No, non l'avete mai fatto. Forse per paura della loro competenza o perché sapete bene che le argomentazioni *pro*-TAV, come minimo, spesso sono delle *fake news*. Sono false. Sono menzogne. motivo è perché l'accordo di base tra Italia e Francia nel 2001 prevedeva, all'articolo 1, che i lavori partissero a saturazione della linea esistente, attualmente sfruttata per meno del 15 per cento. Quindi, questo è il mattone e la base. stanno, allora, questi enormi flussi di merci citati tra noi e Lione? Le proiezioni fatte venti anni fa, di aumento del traffico, sono miseramente crollate, come confermato recentemente dallo stesso Osservatorio della Torino-Lione. Inutile, quindi, far andare un treno merci, non un treno passeggeri, come ho sentito, in gallerie da 57 chilometri alla velocità di 160 chilometri orari, guadagnando, rispetto all'attuale linea, una manciata di minuti. Secondo punto: perché non è mai partita l'opera? Perché, visto che non c'è un solo centimetro del *tunnel* di base di quest'opera? Quest'opera non ha un centimetro di buco. Fino ad oggi sono state realizzate solo attività di riconoscimento geologico, comprese quelle in Francia, perché, più volte, anche la Francia ha fatto un passo indietro. La Corte dei conti francese molto chiaramente - e ho qua il documento ha detto che l'opera è troppo cara e consiglia di ammodernare quella esistente. In più, ha ricordato alla Francia che anche altri Paesi, come Slovenia e Ungheria, hanno preferito migliorare l'esistente, piuttosto che imbarcarsi in opere costosissime e inutili. Più volte l'Europa, che ha decine di progetti ad alta priorità, ha modificato la destinazione dei fondi ad altri Stati membri. Inoltre, persino il Portogallo ha rinunciato all'opera senza pagare un centesimo di penale, pur avendo già

Oggi il traffico di merci avviene prevalentemente sulle direttrici Nord-Sud e non su quelle Est-Ovest. Andate in Svizzera - ne avete parlato anche voi - a dare un'occhiata. Assodato che non ci sono flussi di merci che giustifichino quest'opera e che la linea attuale può portare TIR e *container*

non ci sono penali da pagare.

a qualunque pretesa risarcitoria eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio, nonché a qualunque pretesa anche futura anche futura connessa al mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi». Questo è ribadito anche all'articolo 3 della legge di ratifica 5 gennaio 2017, n. 1, precedentemente richiamata. Identica previsione è contenuta nella delibera del CIPE n. 67 del 2017, nel combinato disposto degli articoli 1 e 6 del deliberato. Io parlo di cose vere, scritte nero su bianco. penali nei rapporti internazionali. Si tratta di decisioni rimesse agli Stati sovrani, come ricorda anche l'Avvocatura dello Stato nella sua relazione giuridica, che devono essere solidamente ancorate alla sostenibilità socio-economica e finanziaria dell'intera opera, secondo le stesse norme europee. Non si vede come possano imputarsi responsabilità gravi in capo agli Stati quando questi presupposti mancano, cioè quando mancano i soldi. Esiste, infine, un precedente. Mi riferisco al Portogallo, che nel 2012 cancellò la propria tratta ad alta velocità Lisbona-Madrid. Non ci fu alcuna richiesta di indennizzo o altra compensazione da parte della Commissione europea e della Spagna. Quindi, nessuna penale, tranne le inutili minacce di TELT e il *diktat* dell'Unione europea. Parliamo dei costi. La linea dovrebbe costare 9,6 miliardi di euro, attualizzati al 31 dicembre 2017, più 1,4 miliardi già spesi tra studi preliminari, indagini, gallerie geognostiche, arriviamo così a oltre 11 miliardi di euro. Considerato che, per adesso, c'è un solo impegno verbale impegno verbale dell'Unione europea per l'incremento del contributo dal 40 al 50 per cento, potremmo anche non ricevere i soldi. Il finanziamento del *tunnel* è di fatto rinviato all'approvazione del bilancio pluriennale dell'Unione europea del 2021 e i fondi già stanziati nel Grant Agreement non potranno essere utilizzati a causa dei ritardi, ma soprattutto perché l'articolo 16 dell'accordo del 2012 impone a Italia e Francia la disponibilità certa del finanziamento di tutta l'opera, compreso l'importo del 40 per cento promesso,

Ma tutto ciò non servirebbe ripeterlo, perché è scritto nero su bianco nell'analisi costi-benefici che l'opera non conviene e non è una *fake news*. Si è impiegato tanto tempo proprio per approfondire adeguatamente la materia. Non dimentichiamo che, per di più, c'è una ripartizione asimmetrica. Oggi è indispensabile che la ripartizione dei costi sia ridiscussa tra Italia e Francia, alla luce del fatto che i due Paesi non vogliono fare più le linee di accesso al *tunnel*. Tale decisione modifica questa ripartizione asimmetrica,

anche il cantiere italiano, se li aggiudicherebbero senza leggi antimafia. Dovranno però aspettare un po', perché sull'intera fattibilità dell'opera, la Francia deciderà nel 2038. Capito? Ma come potete pensare di spendere miliardi per un'opera inutile che, se tutto procede come desiderato dai promotori, potrebbe essere terminata tra trent'anni, quando proprio oggi mi dovete spiegare - lo dico ai lucani presenti - come andrete a Matera, città della cultura 2019? 2019? Questo Paese è stanco di vedere sprecati i soldi. Questo Paese vuole strutture adeguate, muoversi e viaggiare su tratte locali e non andare a lavorare stipati come sardine, in carri bestiame, farsi una gita senza dover prendere due bus e un taxi. TELT non ha alcun titolo o via libera (ancorché silenzio-assenso) al lancio delle gare TAV. Qualora TELT procedesse in tal senso, questo comporterebbe una grave e diretta violazione degli accordi Italia-Francia, che sono legge vigente dello Stato italiano. Il Governo è direttamente responsabile dell'operato di TELT.

TELT. La Commissione europea e l'INEA sono perfettamente a conoscenza di ciò. Anche se TELT non lanciasse lunedì 11 marzo le gare TELT, la Commissione europea vorrebbe decurtare oltre 300 milioni di euro di sovvenzioni assegnate. Ma la Commissione europea non può imporre il calendario. Tale situazione e l'esatta replica di quanto già visto nel 2013 col Governo Monti. Il grave ritardo cui assistiamo è diretta responsabilità di chi doveva agire per tempo e non ha agito, a cominciare dai commissari dei Governi passati. Ho finito, ma prima voglio dirvi una cosa: qui non ci sono solo in gioco miliardi sottratti a scuole, ospedali, ferrovie utili; qui c'è una questione di ordine etico e morale. Lo Stato ha spianato la volontà popolare con la violenza; lo Stato non ha ascoltato i cittadini; lo Stato si è comportato da dittatore calpestando tutto e

Non solo vogliamo mantenere una promessa fatta tanto tempo fa da Beppe e tutti noi, ma li ringrazieremo per quello che hanno fatto per il Paese e soprattutto per l'esempio che ci hanno dato: la sovranità appartiene al popolo e quando il popolo è unito, nessuno può batterlo.

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno

Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante ratifica ed esecuzione di due accordi, rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale, sottoscritti dall'Italia e dalla Bielorussia nel giugno 2011. Mi preme sottolineare che il testo in esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente ai soli due accordi con la Bielorussia, il testo del disegno di legge di ratifica di numerosi trattati internazionali bilaterali proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura, con atto del Senato n. 2812 che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato in data 11 ottobre 2017, senza peraltro poter vedere completato il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura. I due accordi con la Bielorussia oggetto della presente ratifica rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale sono composti ciascuno di 11 articoli e definiscono il quadro giuridico entro cui far continuare e far crescere la collaborazione bilaterale anche attraverso il coinvolgimento della società civile. Il primo dei due accordi è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi internazionali dei due Paesi, in particolare nei settori della ricerca fondamentale ed applicata, della tecnologia industriale e dell'innovazione. Il secondo sulla cooperazione culturale, è a sua volta finalizzato alla realizzazione di programmi di attività comuni per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale, che potranno assumere, tra le altre, le forme dell'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche, della promozione di contatti tra enti ed associazioni culturali, della traduzione di opere letterarie, della intensificazione dei rapporti tra istituzioni museali. Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in circa 170.000 euro annui e in 176.820 euro a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del provvedimento. Evidenzio, per ultimo, come la ratifica degli accordi non presenti profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia, risultando i testi in esame strettamente correlati agli altri strumenti giuridici internazionali dedicati ai temi culturali e scientifici già sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione,

Signor Presidente, con il suo permesso vorrei solamente dichiarare il voto convintamente favorevole del Gruppo Partito Democratico e chiedere di poter lasciare agli atti il testo del mio intervento.

i due accordi con la Bielorussia oggetto della presente ratifica, rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologia e di cooperazione culturale, definiscono il quadro giuridico entro cui far crescere la collaborazione bilaterale e offrono all'Italia l'opportunità di avere un interlocutore privilegiato e un mercato di sbocco importante per i nostri prodotti e servizi. Noi del MoVimento 5 Stelle da sempre siamo favorevoli agli accordi di cooperazione culturale con altri Paesi, perché crediamo che siano le basi per una reciproca conoscenza e collaborazione e permettano la creazione di un contesto favorevole per promuovere il nostro ruolo economico. Credo pure che quando parliamo di mondo della cultura in crisi, in Italia dobbiamo tener conto dell'opportunità di diffondere la nostra cultura, il nostro stile di vita e i nostri prodotti e servizi nel mondo, a partire dalla grande competenza dei nostri Atenei, che - permettetemi di dirlo - sono all'avanguardia. Accordi di questo tipo sono uno strumento privilegiato, al quale dobbiamo ricorrere in maniera ancora più frequente in questa legislatura. Nello specifico, l'accordo di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia permetterà certamente di produrre buoni risultati insieme ai *partner* bielorussi. In particolare, noi siamo tra i primi posti al mondo per ricerca e tecnologia e possiamo cogliere appieno i benefici di questa cooperazione, dando anche ai nostri docenti la possibilità di far conoscere il *know how* italiano all'estero, aumentando così il prestigio dei nostri centri di ricerca. ricerca. Il secondo Accordo sulla cooperazione culturale permetterà di dare vita a collaborazioni proficue e a nuove forme dell'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche, della promozione di contatti tra enti e associazioni culturali, culturali, della traduzione di opere letterarie e dell'intensificazione dei rapporti fra istituzioni museali. Mi sembra molto interessante, poi, il richiamo alla tutela del patrimonio culturale, che potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni future anche in campo economico. Signor Presidente, ci auguriamo che possano aumentare le opportunità di collaborazione con il popolo bielorusso, ma soprattutto che la via della promozione del nostro ruolo culturale e scientifico diventi uno degli strumenti della nostra cooperazione internazionale, anche in considerazione della nostra grande esperienza. Mi permetto di dire, in conclusione, che la cooperazione culturale con altri popoli va vista sempre come un ponte, una mano tesa alla società con cui ci relazioniamo, ancor prima di un accordo con questo o quel Governo. Lo dico perché è importante comprendere il nostro ruolo internazionale, che non può più essere quello del passato. In questo nuovo contesto multipolare, l'Italia deve essere protagonista della mediazione, deve promuovere la pace e il benessere e proporsi nello scambio di conoscenze e nella tutela del patrimonio umano in tutte le sue forme. Per questo il Parlamento, nell'espletamento del suo lavoro, deve essere scevro da pregiudizi e pragmatico nell'agire, avendo sempre a cuore l'interesse del nostro Paese. Facendo ciò, dobbiamo inevitabilmente valorizzare le nostre peculiarità; e la promozione della cultura e della ricerca è una di queste. Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato su questa ratifica. *(Applausi

sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica di Corea rispettivamente nell'ottobre 2005 e nel febbraio 2007. Come si evince dalla relazione introduttiva, il testo al nostro esame ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente ai soli due Accordi con la Corea del Sud, l'atto Senato n. 2813, recante ratifica di numerosi accordi internazionali bilaterali, che, presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato il 28 giugno 2017, ma non poté vedere completato il proprio *iter* parlamentare a causa della fine della legislatura. Gli Accordi in via di ratifica sono finalizzati a definire la cornice giuridica entro cui far crescere la già ottima collaborazione fra l'Italia e la Corea del Sud nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia. In particolare, con il primo dei due testi, quello sulla cooperazione culturale, le parti esprimono il comune auspicio a voler promuovere la cooperazione bilaterale e multilaterale nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale e archeologico, dei giovani e dello sport (articoli 1 e 2). che verte sulla cooperazione scientifica e tecnologica, si mira a superare un precedente trattato bilaterale di settore, risalente al 1984, e a promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse (articolo 1), sia sul piano bilaterale, in particolare mediante la stipula di specifici accordi tra Ministeri, istituzioni, università e centri di ricerca coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica (articolo 2), che su quello multilaterale (articolo 3). Gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati complessivamente in circa 790.000 euro annui e e in 815.170 euro a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del provvedimento. Evidenzio, da ultimo, come la ratifica degli accordi non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia, risultando i testi in esame strettamente correlati agli altri strumenti giuridici internazionali dedicati ai temi culturali e scientifici già sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

di collaborazione scientifica e tecnologica tra la Corea del Sud e l'Italia sono ottimi e penso che questo Accordo ci aiuti a svilupparli ancora di più. In particolare, la cooperazione culturale ci permetterà nuove forme di scambio nel settore delle arti e della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale e archeologico, dei giovani e dello sport. Per ciò che riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica, penso che vada sottolineato che la Corea è oggi uno dei *leader* mondiali in questo settore e quindi è grande l'attenzione che il Governo coreano dà agli investimenti e alla ricerca sull'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di far parte dei dieci Paesi *leader* in tale ambito. Penso che sia importante che l'Italia, che intende porsi in una posizione importante in estremo Oriente, profilandosi sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati *partner* particolarmente avanzati,

Signor Presidente, colleghi, colleghe, signori rappresentanti del Governo, come ben sapete i rapporti tra il nostro Paese e la Repubblica della Corea del Sud sono ormai consolidati da almeno Il primo Accordo fu firmato a Seul nel lontano 1965. Con il passare degli anni l'iniziativa diplomatica tra i due Paesi si è intensificata sempre di più e gli Accordi e i Protocolli di intesa sono stati man mano aggiornati e modellati rispetto alle esigenze dei firmatari. Del resto, se analizziamo i dati storici della Corea del Sud non possiamo che constatare la progressiva crescita economica e demografica di quel Paese: nel 1965, anno del primo accordo, la Corea del Sud contava 28 milioni di abitanti; oggi ne conta 50 milioni. Sempre nel 1965 il reddito *pro capite* era di 79 dollari statunitensi; oggi è di 31.000. La crescita del PIL è stata costante con punte del 4 per cento annuale. Gli Accordi oggetto oggi di ratifica vanno a definire un quadro giuridico nel quale si estrinseca la potenzialità dei rispettivi Paesi. Il primo accordo riguarda la promozione e cooperazione bilaterale e multilaterale attinente alla cultura, all'istruzione e al patrimonio culturale e archeologico. È inutile che vi descriva l'interesse di quel popolo per l'Italia, per le nostre arti e la nostra cultura. Appare persino superfluo elencare i dati delle presenze turistiche di visitatori sudcoreani in Italia: vi posso assicurare che si attestano tra i più significativi del continente asiatico e sono in costante crescita. Lo scambio culturale nel campo musicale si è concretizzato nella presenza stabile del padiglione della biennale di Venezia interamente dedicato al Paese asiatico.

L'interesse dei coreani per il Paese del bel canto si appalesa nelle selezioni per i corsi di canto. Tanto per renderci conto di cosa parliamo, è doveroso citare alcuni dati: nel 1997 nel conservatorio di Santa Cecilia a Roma, su 30 candidati ammessi, tra i 180 che avevano presentato domanda, 23 erano ragazzi coreani. Inoltre, secondo gli ultimi dati raccolti, sembrerebbe che siano quasi 3 milioni i giovani coreani impegnati nei conservatori e nelle scuole di musica occidentali. Sono numeri impressionanti che ci fanno capire l'importanza di questo accordo. Il secondo accordo, che di fatto supera il precedente del 1984, si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo del partenariato scientifico e tecnologico attraverso accordi tra Ministeri, università e centri di ricerca. Ricordiamo che anche su questo versante l'interscambio bilaterale ha raggiunto complessivamente i 10 miliardi e 800 milioni di dollari, con un avanzo commerciale a noi favorevole di circa un miliardo e 800 milioni di dollari. Basterebbero questi dati a giustificare l'interesse reciproco alla ratifica e all'esecuzione dei citati accordi. Vi chiedo pertanto di votare favorevolmente al disegno di legge n. 678 per la ratifica degli Accordi tra l'Italia e la Repubblica della Corea

relazione. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo del giugno 2017 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO). Ricordo che è l'organizzazione che promuove lo Stato di diritto e le pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo e in situazioni postbelliche. Il testo in via di ratifica è importante perché consolida la presenza in Italia della sede dell'IDLO, scongiurando il rischio di un suo possibile trasferimento all'estero.

in oggetto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Per i motivi che ho brevemente riassunto, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. **Saluto

paese che conosco, per esserci stato. Grazie della vostra visita.

è un'organizzazione intergovernativa che si dedica alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, in transizione economica e nei Paesi in situazioni postbelliche. giustizia. Il lavoro svolto dall'Organizzazione integra anche le attività di altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma, che operano nel campo della sicurezza alimentare e dello sviluppo dell'agricoltura sostenibile.

L'IDLO è un'organizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello Stato di diritto e delle pratiche di buon governo nei Paesi in via di sviluppo, in transizione economica e nei Paesi reduci da conflitti armati. Va inoltre ricordato che ha lo *status* di osservatore presso la sede delle Nazioni Unite a New York e partecipa costantemente a *meeting* che riguardano i temi da essa trattati; lo fa attraverso la formazione di giuristi, la produzione di documenti analitici e la promozione del dibattito sull'accesso alla giustizia, sul diritto dei minori, sullo sviluppo sostenibile, sulla pace e la democrazia, sulla salute e sulle riforme legali in 47 Paesi. L'IDLO produce studi, consulenze e alta formazione, con l'intento di migliorare il quadro giuridico dei Paesi poveri o in via di sviluppo, armonizzandolo con quello dei Paesi ricchi o industrializzati aderenti all'organizzazione. Dai lavori dell'IDLO molti Governi prendono spunto per riforme della giustizia o per interventi normativi sui temi trattati dall'Organizzazione. È il caso di citare l'intervento dell'Organizzazione in Guatemala, a tutela dei diritti degli indigeni. Nel 2014 l'IDLO ha formulato una serie di raccomandazioni specifiche al Governo per aiutarlo a rafforzare le istituzioni e per ridurre i conflitti legati alla terra nelle aree rurali, sostenendo una proposta di aumento dei finanziamenti governativi per attuare progetti di sviluppo sostenibile. L'Organizzazione promuove inoltre il ruolo delle donne nella giustizia e l'adozione di provvedimenti per mitigare le cause della disparità di genere, soprattutto in Africa, attraverso un *report* analitico con una serie di esperienze che hanno migliorato l'accesso delle donne alle carriere nel settore della giustizia. Con il voto di oggi manteniamo aperto uno spazio importantissimo che si traduce anche in maggiori opportunità per i nostri giuristi di potersi confrontare con un ampio panorama internazionale direttamente a Roma. Il MoVimento 5 Stelle è da sempre una forza politica attenta al mondo della ricerca, sia tecnico scientifica che di altra natura, perché possiamo valorizzare il nostro patrimonio più grande: i nostri ricercatori, i nostri docenti, la nostra scuola pubblica ed evitare che i nostri giovani vadano all'estero a cercare opportunità. Noi dobbiamo invece creare le condizioni, che sono ovviamente molteplici, perché non solo i centri di ricerca scientifica, ma anche le organizzazioni come l'IDLO, possano vedere nell'Italia un centro culturale stimolante a livello mondiale.

***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018***

consapevole che i lavori di ratifica che arrivano in Assemblea e che vengono sovrapposti uno all'altro generano un minimo di confusione. Devo però ringraziare anzitutto gli esponenti del Governo che hanno assunto lo stesso atteggiamento che ha avuto il vice ministro Del Re, ascoltando con grande attenzione e pazienza quattro ratifiche svolte velocemente. Ringrazio tutti i colleghi per la loro collaborazione. Faccio solo un appunto. A nome di tutta la Commissione, quale Presidente della Commissione affari esteri, devo sottolineare che è veramente poco piacevole nel momento in cui chi deve fare dichiarazioni di voto o svolgere la relazione di introduzione a un provvedimento, con la dignità di qualsiasi altro componente di Commissione, si prende il tempo necessario, ascoltare mormorii quando i tempi sulla discussione delle ratifiche vanno oltre quello che qualcuno in Assemblea considera necessario. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto)*. Lo dico con grande franchezza, ringrazio tutti i colleghi e spero che non accada più. Mi assumo tutta la responsabilità di questa dichiarazione perché la Commissione affari esteri, anche se svolge velocemente

siamo grati a chi ci ha preceduto per aver permesso, nella storia del nostro territorio, di accogliere

fruiscono di questa scuola di altissima formazione, che costituisce un *unicum* mondiale a questo livello; sono più di 70 i docenti e, all'interno del percorso di formazione, si avvicenda un numero ancora superiore di personaggi che, con seminari ed eventi particolari,

che ha come obiettivo l'attivazione di percorsi di ricerca e di formazione su temi importanti della *governance* globale, quali la democrazia, i diritti, la finanza, il commercio, i cambiamenti climatici e la diplomazia; tutti temi che sono

facendo riferimento a quello che ho detto poco fa, ovvero al fatto che tutti noi dovremmo guardare con interesse all'Istituto universitario europeo.

differentemente da quanto sembrerebbe emergere in uno dei due atti di sindacato ispettivo in parola, questo Ministero, unitamente agli altri soggetti istituzionali, ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole, cercando di garantire tutte le varie realtà e differenti sensibilità, nell'interesse esclusivo di studenti, famiglie e di tutte le componenti del mondo della scuola. Terzietà, imparzialità ed equità sono i princìpi che hanno, infatti, sempre improntato le scelte e le azioni poste in essere da questo Ministero. Tuttavia, è necessario premettere che il questionario sul bullismo omofobico, oggetto delle interrogazioni parlamentari, trova fondamento in un accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di analisi, studio, ricerca, formazione e sperimentazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo omofobico, sottoscritto nel novembre 2017 tra la Regione Umbria, l'Università degli studi di Perugia, l'Ufficio scolastico regionale, l'Ufficio per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Umbria e L'impegno dell'Ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'accordo in argomento, è stato volto ad agevolare e sostenere la diffusione di informazioni nelle scuole per lo svolgimento dell'attività di ricerca. È per questo motivo che lo stesso Ufficio scolastico regionale ha informato le istituzioni scolastiche della Regione - selezionate mediante sorteggio pubblico, al fine di individuare le 54 classi campione dell'avvio della ricerca in questione, precisando che le stesse sarebbero state libere di non aderirvi. La procedura prevista ha consentito il trasparente coinvolgimento tanto delle comunità scolastiche interessate, attraverso l'approvazione da parte degli organi collegiali dell'adesione alla ricerca, quanto delle famiglie, attraverso l'acquisizione del consenso scritto alla somministrazione e compilazione da parte dei propri figli del questionario. Difatti, l'Università degli studi di Perugia, al momento del contatto con le istituzioni scolastiche interessate, ha trasmesso, unitamente al predetto questionario, il modulo di acquisizione del consenso da parte dei genitori. Secondo quanto riportato nella relazione pervenuta a questo Ministero dall'Ufficio scolastico interessato, tale meccanismo di libertà di scelta ha fatto sì che più del 60 per cento delle scuole contattate abbia deciso di non partecipare alla ricerca. È di tutta evidenza, dunque, che le scuole hanno lavorato in piena collaborazione con le famiglie, recependo le istanze provenienti da queste e preoccupandosi di tutelare pienamente l'interesse dei minori. Non è un caso, difatti, che la nota con la quale l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato l'avvio della ricerca abbia evidenziato l'assenza di vincoli e la necessità di valutare l'opportunità della partecipazione, in considerazione del contesto scolastico e delle osservazioni degli organi collegiali e dei genitori; valutazione che, come dimostra il numero definitivo delle scuole aderenti alla ricerca, è avvenuta. È doveroso ricordare che, sempre secondo quanto riportato nella sopra richiamata relazione, è stata proprio la direzione scientifica della ricerca dell'Università degli studi di Perugia ad aver selezionato dalla letteratura scientifica internazionale il questionario e ad averlo inviato alle istituzioni scolastiche, senza aver sottoposto lo stesso al vaglio dell'Ufficio scolastico regionale. Ad ogni modo, quest'ultimo non appena è venuto a conoscenza del questionario, tenuto conto che lo stesso non era stato condiviso e considerato l'impatto che il medesimo aveva avuto nel contesto scolastico regionale, ha proceduto formalmente a chiedere all'Università degli studi di Perugia e alla Regione Umbria di rivedere la formulazione dei questionari e le modalità di realizzazione del progetto, sospendendo, di fatto, l'operazione di avvio alla somministrazione del questionario. in una comunicazione di chiarimento inviata dall'Università degli studi di Perugia all'Ufficio scolastico regionale, si precisava che il questionario in oggetto, al momento del clamore mediatico, non era ancora definitivo, in quanto, a seguito di osservazioni e suggerimenti provenienti prevalentemente da dirigenti scolastici che lo avevano letto, si stava procedendo ad alcune modifiche, tra le quali, per l'appunto, l'eliminazione della parte di questionario destinato alla scuola secondaria di primo grado, contenente domande relative all'orientamento sessuale, all'orientamento religioso e all'orientamento politico. Si evidenzia, infine, così come riportato nella relazione dell'Ufficio scolastico regionale, che il *link* definitivo per la somministrazione del questionario non è stato mai inviato a nessuno e la somministrazione del questionario non è mai iniziata in alcuna istituzione scolastica. Stante tale situazione, nel dicembre 2018 l'Ufficio scolastico regionale ha ritenuto opportuno informare il Ministro della richiesta di riformulazione dei questionari e di revisione delle modalità di realizzazione del progetto, con conseguente sospensione della ricerca. Successivamente, il ministro Bussetti ha reso pubblica la sospensione dei questionari, ritenendo necessario un approfondimento e chiedendo, altresì, di rivederne la formulazione degli stessi e di cambiare le modalità di realizzazione del progetto. In aggiunta a quanto sopra rappresentato, occorre sottolineare che la mancata adesione da parte di più del 60 per cento delle scuole coinvolte non avrebbe consentito il reclutamento del campione necessario, facendo venir meno la rappresentatività delle classi. I risultati ottenibili, secondo i numeri registrati, sarebbero stati, pertanto, non corrispondenti alla realtà del territorio e poco utili all'analisi del fenomeno in oggetto. In questo scenario, è doveroso rimarcare come il MIUR sia da tempo impegnato sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (come prevede la legge n. 71 del 2017) e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non riconducibili solo al contesto scolastico. In particolare: Generazioni Connesse, il tavolo tecnico interministeriale e il progetto Piattaforma Elisa. In conclusione, trattasi di strumenti fondamentali in quanto solo la formazione nei giovani di una cultura fondata

Signor Presidente, ringrazio il collega Sottosegretario del Governo, che ritiene di aver salvato qualche bambino bullizzato con la sua triste replica, totalmente burocratica, piena di parole senza senso che non aiutano. Non stiamo parlando, caro Sottosegretario del Governo, di pezzi di carta, di delibere, di atti. Stiamo parlando della vita di molti ragazzini presenti nelle nostre scuole. Le segnalo «la Repubblica» di oggi, dove si legge che una ragazzina non è stata solo bullizzata, ma violentata violentata dal padre e segregata in casa, perché si vergogna di avere una figlia lesbica. Se lei pensa di aver dato una risposta esaustiva con la sua nota, la invito a uscire dal Palazzo e a andare a vedere quello che accade nelle scuole, nei nostri quartieri, nelle nostre città, dove ormai, purtroppo, per la immensa diffusione di odio continua, che viene fatta anche, purtroppo, a elevatissimi livelli delle nostre istituzioni, ogni diversità è considerata da punire; ogni diversità è considerata una vergogna; ogni ragazzino, semplicemente perché indossa una maglietta rosa ed è un maschio, va in qualche modo preso di mira. È su questo che io io ho presentato l'interrogazione, insieme ai miei colleghi umbri, la senatrice Ginetti e il senatore Grimani. È su questo che la scuola interviene nel diventare

la legge contro l'omofobia. Il punto vero è proprio questo. Mettiamo l'omofobia sullo stesso piano di tutte le altre violenze, come il femminicidio e tutti i reati contro la persona,

sia presente sul volantino. In quella grande manifestazione delle famiglie del mondo sono presenti persone che, nel loro Paese, ritengono che vada data la pena di morte - o chissà

Signor Presidente, colgo l'occasione per ringraziare le associazioni dei genitori che hanno denunciato l'abuso che si stava perpetrando nelle scuole umbre, segnalando tempestivamente

ratificata dal nostro Paese, stabilisce che lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Quest'alleanza educativa tra la famiglia e la scuola

come utilizzare i propri organi genitali. Allora se, secondo il Partito Democratico, questa è lotta al bullismo, noi siamo convinti che questo sia l'esatto contrario: questo è bullismo sui minori bullismo di pochi invasati che con i nostri figli vogliono fare i loro esperimenti sociali del tutto inaccettabili. I fatti sono duri da smentire e, quindi, andiamo a prendere il questionario che si stava somministrando ai nostri figli e leggiamo che cosa c'era scritto. Costringere una ragazzina di dieci anni a scegliere se definirsi «esclusivamente eterosessuale», oppure «prevalentemente eterosessuale», oppure «bisessuale», oppure «prevalentemente omosessuale», oppure «esclusivamente omosessuale» oppure «asessuale», è qualche cosa di vomitevole. È una vergogna che qualcuno pensi di poter indottrinare i nostri figli in questo modo inaccettabile. Come del resto è una vergogna che quei minori siano costretti, nella mente di qualche ricercatore, ad associare tale domanda ad altre due contigue legate al proprio sentimento religioso: «quanto consideri importante la religione nella tua vita»; e al proprio orientamento politico: «ti definisci di estrema sinistra, di sinistra, di centrosinistra, di centro, di centrodestra, di destra o di estrema destra»? Questo su un bambino di dieci anni è qualche cosa di scandaloso. Altro che educazione contro l'omofobia! Questo è indottrinamento politico-ideologico. *(Applausi Lo dico con estrema chiarezza ai senatori del Partito Democratico: finché ci saremo noi, queste porcherie non saranno date ai nostri figli. *(Applausi dal coinvolgendo le famiglie e non contro le famiglie; si fa educando i figli al rispetto del corpo e non sessualizzandoli precocemente; si fa usando il buonsenso e non sciocche ricerche infarcite di ideologia vomitevole. Per fare tutto questo c'è uno strumento che la legge prevede e che il Ministero ha recentemente ribadito in modo autorevole.

e di decidere legittimamente se quei contenuti sono ritenuti o meno adeguati per i propri minori. Ma se il consenso informato è la roba che è stata somministrata ai genitori umbri, nella quale si legge: «Io sottoscritto», «in qualità di genitore di», «frequentante la classe, sezione», «con la presente acconsento alla partecipazione di mio figlio o mia figlia all'indagine attraverso la risposta al questionario», non informa un bel niente. Questo non è un consenso informato, ma è una presa in giro, un prendere i genitori e raccontargli la storia dell'orso. i genitori non accettano più questo tipo di soprusi. Abbiamo sentinelle in tutta Italia, in piedi, sedute. Qualunque tipo di sopruso sarà denunciato, segnalato, intercettato, bloccato. Invito la senatrice Cirinnà, il Presidente e tutti i presenti in quest'Aula a venire alla festa della famiglia di Verona: non sarà la festa dell'odio, ma sarà la festa della famiglia *(Applausi dal

recata dal decreto legislativo n. 216 del 2017, richiamando dichiarazioni che il Ministro della giustizia avrebbe reso a margine della proroga in discussione - quali ad esempio Possiamo dire che ogni volta che uno del PD veniva ascoltato dai cittadini, il PD tagliava la linea, le comunicazioni (...) La norma che abbiamo bloccato, ripeto, ledeva tutti i diritti in gioco: la possibilità innanzitutto di portare avanti le indagini, dando alla polizia giudiziaria la possibilità di scegliere quali intercettazioni fossero rilevanti e quali no, un'attività che deve spettare al pm ma che in questo caso veniva tagliato fuori» chiedono di sapere di quali informazioni il Ministro sia in possesso per affermare che «ogni volta che qualcuno del PD veniva ascoltato, c'era il PD che cercava di tagliare la linea e le comunicazioni», sulla base di quale legge dello Stato, con quali modalità e con quali finalità abbia ottenuto queste informazioni e se non ritenga doveroso, vista la gravità dei fatti riportati, informare subito il Parlamento, se non ritenga che le sue affermazioni siano state gravemente lesive delle prerogative e dei compiti della magistratura e della Polizia giudiziaria e se non ritenga che, nel suo ruolo di Ministro della giustizia, sia tenuto al rispetto dell'applicazione delle leggi vigenti. Nella presente sede, non possono che essere ribadite le medesime considerazioni già svolte in questa stessa Aula lo scorso mese di agosto su un *question time* di analogo tenore. In coerenza rispetto a quanto affermato dal Ministro della giustizia anche nella precedente veste di rappresentante del MoVimento 5 Stelle, occorre preliminarmente riconoscere l'importante ruolo dei *mass media* nella dialettica democratica per la maturazione di una cittadinanza attiva e consapevole rispetto alle vicende politiche del nostro Paese, fermo restando il pieno rispetto delle prerogative della magistratura. Si tratta di un logico quanto elementare corollario del principio costituzionalmente garantito della libera manifestazione del pensiero. Partendo da tali premesse, corre l'obbligo di precisare che le dichiarazioni a cui fa riferimento l'atto di sindacato ispettivo derivano non dalla disponibilità di informazioni riservate da parte di questo Ministro, ma da una attenta osservazione dell'*iter* parlamentare sul disegno di legge di riforma del processo penale contenente anche la delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di pubblicazione delle intercettazioni. Giova, infatti, ricordare la singolare accelerazione dei lavori parlamentari sul citato provvedimento e invero il disegno di legge veniva approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014 e veniva trasmesso alla Camera dei deputati solo il 23 dicembre 2014, oltre quattro mesi dopo e all'indomani degli arresti eseguiti nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, nella quale era emerso il coinvolgimento di taluni esponenti del Partito Democratico romano. Dopo circa sei mesi, il 25 luglio 2015, in una seduta notturna della Commissione giustizia della Camera, veniva approvato l'ormai noto emendamento Pagano relativo al diritto di diffusione di riprese e registrazioni di conversazioni tra privati, laddove, tra le cause di esclusione della punibilità, non veniva ricompreso l'esercizio del diritto di cronaca,; emendamento, questo, poi opportunamente modificato nella versione definitiva in ragione delle allarmanti ricadute sulla libertà di stampa. seduta notturna era stata valutata dall'allora maggioranza indispensabile per una pronta trasmissione in Aula del testo. Difatti, il successivo 27 luglio 2015, il testo del disegno di legge arrivava in Aula della Camera per la discussione, il tutto pochi giorni dopo la pubblicazione su «il Fatto Quotidiano» della nota conversazione tra l'allora *Premier* Matteo Renzi e il comandante interregionale della Guardia di finanza Michele Adinolfi, acquisita nell'ambito delle indagini della procura di Napoli sulla vicenda CPL Concordia, nonché all'indomani della pubblicazione su «l'Espresso» della conversazione tra l'allora governatore della Sicilia Rosario Crocetta e il medico Matteo Tutino. Ancora, il 19 maggio 2017, all'indomani della pubblicazione della conversazione sempre tra l'allora *premier* e suo padre, nell'ambito della vicenda Consip, fu proprio il precedente guardasigilli, l'onorevole Andrea Orlando, a segnalare l'opportunità di procedere all'approvazione del disegno di legge al precipuo scopo di scongiurare tali propalazioni giornalistiche. Pertanto, quelle dichiarazioni nascono, all'evidenza, dalla singolare coincidenza tra l'emersione di vicende giudiziarie che vedevano coinvolti esponenti del Partito Democratico e l'improvvisa accelerazione dell'*iter* parlamentare. L'approccio del Ministero della giustizia verso la materia delle intercettazioni parte dal riconoscimento del ruolo centrale e ineludibile che questo mezzo di ricerca della prova riveste nell'ambito delle indagini. Proprio per tale ragione, il Ministro della giustizia, nell'ottica del confronto che ne contraddistingue da sempre l'operato, ha inteso curare una apposita interlocuzione con tutti gli uffici requirenti del territorio, da cui sono emerse varie criticità della riforma che non possono essere ignorate e che impongono tuttora una riflessione approfondita sulle ricadute che ne discendono. In questa direzione, si iscrive il cosiddetto decreto milleproroghe, con cui si è procrastinata ulteriormente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 216 così da riservare un congruo *spatium deliberandi* nel cui ambito ricercare, in prospettiva migliorativa, un'ottimale declinazione degli equilibri fra garanzie difensive ed efficienza investigativa. La decisione, infatti, risponde alla necessità di riconsiderare l'impianto complessivo della riforma, con l'obiettivo di trovare un giusto ed equilibrato contemperamento tra esigenze parimenti prioritarie, cioè l'efficienza delle indagini, la corretta distribuzione delle funzioni istituzionali tra pubblico ministero e Polizia giudiziaria e la piena tutela del diritto di difesa.

che lo stesso onorevole Bonafede ricopre ancora a tutt'oggi, in qualità di Ministro della giustizia, quanto dell'Assemblea, delle forze politiche e direi addirittura del sistema istituzionale di questo Paese. Lei, signor Sottosegretario, oggi si permette di avallare e difendere le dichiarazioni del ministro Bonafede facendo riferimento a singolari

solo in cinque minuti, avrei modo di riferire a quest'Assemblea quante singolari coincidenze ci siamo trovati ad affrontare dall'inizio della legislatura ad oggi, rispetto a provvedimenti che ci avete portato. Lei però parla di singolari coincidenze rispetto ad affermazioni gravissime rilasciate

singolari coincidenze mi sembrano veramente poco per lanciare accuse di questo tipo, dato che oggi non ci avete portato alcuna ragione o motivazione valida: del resto, se ne aveste avute, immaginiamo che probabilmente avreste agito diversamente, come il vostro dovere istituzionale vi avrebbe imposto. Capiamo che per voi il dovere istituzionale istituzionale sia qualcosa di lontano da quello che concepite, ma probabilmente, se aveste avuto fatti dalla vostra, avreste dovuto fare ben altro. Non avete dunque tali fatti - oggi infatti non siete venuti a raccontarceli - in base ai quali

competenza e il rigore propri di un magistrato si può decidere che uso fare, nel corso di un'indagine, di un giudizio e di un processo, delle dichiarazioni rilasciate da un politico. Non sono i cittadini a dover ascoltare quelle intercettazioni. Di questo noi chiedevamo conto al ministro Bonafede, solo di questo. Lei oggi, ancora una volta, ha perso l'occasione per dimostrare non solo che voi avete il senso delle istituzioni ma che un Ministro della giustizia, prima di rendere dichiarazioni di un certo tipo, deve rendersi conto della delicatezza del suo ruolo e della sua funzione. Avete perso l'occasione per dimostrarci che lavorate nell'interesse del Paese e non solo della vostra propaganda.

come casa mandamentale e destinato in un primo momento a ospitare solo detenuti tossicodipendenti provenienti da altri istituti, riconosciuto nel 2000 come istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti e poi divenuto, a partire dal 2008, luogo per la detenzione anche di detenuti comuni) evidenziando in particolare il sovraffollamento della popolazione ristretta (che conta 68 unità rispetto ai 58 posti disponibili) e la mancanza di 9 unità di personale di polizia penitenziaria (composto da 25 unità effettive su 31 formalmente assegnate, a fronte delle 79 unità in dotazione all'atto dell'apertura della struttura) chiedono di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga urgente intervenire per sanare la condizione di carenza strutturata di organico causata dai tagli lineari della cosiddetta riforma Madia, anche al fine di ristabilire normali condizioni di lavoro, con la riattivazione di posti di servizio essenziali, garantendo adeguata sicurezza all'istituto. Per quanto attiene alla dotazione organica, risulta che presso l'istituto di Giarre sono effettivamente in servizio, al netto dei distacchi in entrata e in uscita,

L'unica carenza viene registrata nel ruolo dei sovrintendenti, rispetto a cui manca una delle quattro unità previste. Si tratta, all'evidenza, di un margine di scopertura che, se debitamente correlato al contesto dell'intero territorio nazionale, può definirsi modesto. A contenerne la criticità, del resto, converge anche il dato relativo alla popolazione carceraria, in quanto alla data dello scorso 7 gennaio erano presenti presso la struttura di Giarre 62 detenuti rispetto ai 58 previsti, venendo in rilievo un tasso di sovraffollamento nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 126 per cento circa. Peraltro, il rapporto complessivo tra Corpo di polizia penitenziaria e detenuti si attesta su una percentuale del 56,5 per cento, come tale in linea con la media nazionale. Ad ogni buon conto, tra le priorità del Ministero della giustizia rientrano le iniziative volte a rafforzare il contingente della Polizia penitenziaria e a ripristinare conseguentemente condizioni di maggior sicurezza nelle carceri italiane. In questa direzione si iscrive il significativo stanziamento di risorse pari a 71,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021, previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e con cui è stata pianificata l'assunzione di 1.300 unità del Corpo di polizia penitenziaria nell'anno 2019 e di 577 unità nel periodo 2020-2023, proprio al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche tenuto conto delle indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario. Inoltre, è prevista l'immissione in ruolo di 976 allievi vice ispettori, che hanno frequentato il corso di formazione appena concluso. Quanto invece al ruolo dei sovrintendenti, sono tuttora in corso le procedure per il concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo. Peraltro, proprio con riferimento alla dotazione organica della casa circondariale di Giarre, va detto che la stessa ha fruito del recente incremento di due unità maschili nel ruolo di agenti-assistenti, tramite mobilità ordinaria collegata all'immissione in ruolo degli allievi

ANASTASI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il signor Sottosegretario per la risposta. La Provincia di Catania attendeva da molto tempo questo tipo di interessamento. casa circondariale di Giarre, infatti, è stata oggetto in passato di più interrogazioni parlamentari, ma purtroppo i Governi precedenti non sono mai stati all'altezza di dare una risposta, né verbale, né fattiva. Mi corre l'obbligo di ricordare che, appena un anno fa, alcune sigle sindacali hanno protestato presso la prefettura di Catania, denunciando le condizioni di lavoro degli agenti della polizia penitenziaria costretti a turni massacranti, con rischio anche per la stessa sicurezza della casa circondariale. Per effetto dei tagli dovuti in particolare alla legge Madia, che hanno ridotto gli agenti prima da 44 a 39 e poi fino a 34,

Basti pensare che il box di accesso alla casa circondariale è spesso sguarnito e il cancello deve essere tenuto necessariamente chiuso, perché nessuno può controllare i movimenti in entrata e in uscita. non si può pensare neppure di svolgere altri servizi, quali per esempio gli accompagnamenti: così, quando un detenuto deve essere accompagnato presso l'ospedale, che dista 30 chilometri, o presso il tribunale, che è altrettanto lontano, deve essere distaccata un'unità da un'altra casa circondariale. Queste unità devono venire a Giarre, devono prendere il detenuto, lo devono accompagnare di nuovo a Catania, poi devono riaccompagnarlo a Giarre e tornare di nuovo a Catania, quindi con uno spreco enorme

anche come «boschetto di Rogoredo», limitrofa all'omonima stazione ferroviaria e ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti, è costantemente attenzionata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza e dalle Forze dell'ordine. Il degrado e le condizioni di precaria sicurezza di quell'area sono state, peraltro, oggetto di una seduta *ad hoc* del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto nell'autunno scorso dal Ministro dell'interno, che ha confermato l'impegno per una più incisiva attività di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree del parco, allo scopo di addivenire ad una risoluzione definitiva della problematica, assicurando, altresì, il pieno sostegno a specifiche progettualità del Comune di Milano. Gli impegni assunti in quella sede si sono tradotti in una serie di iniziative che si muovono su tre direttrici fondamentali: la riqualificazione urbana e ambientale dell'area, la profilassi sanitaria e il rafforzamento dell'attività di prevenzione e contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Sotto il primo aspetto, si informa che la società Rete ferroviaria italiana (RFI) ha completato già nel mese di settembre del 2018 la costruzione presso la stazione ferroviaria di Milano-Rogoredo di un muro in cemento armato lungo 600 metri per evitare i continui scavalchi e gli indebiti attraversamenti dei binari, oltre ad aver eseguito opere di tamponatura degli accessi. La stessa società ha inoltre programmato la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza per un totale di 85 telecamere, il cui inizio dei lavori è previsto entro l'anno in corso. Analogo sistema di controllo sarà realizzato anche nelle stazioni di Lambrate, Greco Pirelli, Porta Garibaldi e nella stazione di Pavia. Ulteriori iniziative di riqualificazione economica e sociale dell'area vedono il coinvolgimento attivo di Regione, Comune e forze di polizia per l'avvio in tempi rapidi di un progetto di recupero urbanistico incentrato sulla realizzazione nell'area in in questione del Palazzo del ghiaccio, in vista dell'eventuale assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina. Nella stessa direzione si segnala la possibile realizzazione di un progetto per il trasferimento della sede della fondazione Exodus all'interno del parco. Sotto il profilo sanitario invece, è stato già programmato l'avvio di uno specifico progetto - elaborato tra Regione Lombardia d'intesa con il Comune di Milano e con il coinvolgimento del privato sociale - per disincentivare il consumo di droga, ridurre il danno per gli assuntori abituali e garantire immediati soccorsi sul posto. Il previsto aumento del numero di giornate e dei tempi di presenza degli operatori sanitari sul posto consentirà anche di intensificare l'approccio mirato ai consumatori occasionali, con particolare riguardo ai minori. Per quanto riguarda il più specifico versante del contrasto allo spaccio di stupefacenti, si evidenza che nell'area in questione siano costanti già da tempo i controlli quotidianamente assicurati dalle Forze dell'ordine. Numerose sono state le operazioni di polizia che hanno portato all'elevazione di sanzioni amministrative e al sequestro di sostanze stupefacenti, oltre all'adozione di provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti degli assuntori non residenti. In particolare, nell'ultimo trimestre sono state controllate nella zona circa 1.000 persone. Tale attività, condotta dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla polizia locale - che colgo l'occasione per ringraziare - ha avuto i seguenti esiti: 24 persone arrestate, 45 denunciate, 90 segnalate per l'applicazione dei provvedimenti di foglio di via obbligatorio da parte dell'autorità di pubblica sicurezza; circa 800 veicoli controllati; circa 3 chili di sostanze stupefacenti sequestrate. Infine, quanto all'auspicata attivazione di un presidio permanente della polizia ferroviaria nella stazione di Milano Rogoredo, si informa che il Dipartimento della pubblica sicurezza, rivalutando i motivi che avevano portato nel 2004 alla sua chiusura, ha deciso di ripristinarlo prevedendo un organico di 18 dipendenti. A tal fine, sono già stati individuati i locali che ospiteranno il nuovo presidio e avviate le procedure per la realizzazione dei necessari interventi strutturali. Nelle more delle istituzioni del nuovo reparto, comunque, l'organico della Polfer di Milano-Lambrate - che dal 2004 ha assorbito la competenza territoriale sullo scalo di Rogoredo - è stato già potenziato con l'assegnazione di due unità che si sono recentemente aggiunte all'organico effettivo, ora pari a 35 unità, con ciò consentendo un aumento dei controlli con riferimento

di cui questa interrogazione è stata un elemento perché è da tempo che, anche con diversi interventi di fine seduta, insistiamo perché ci sia un intervento al boschetto di Rogoredo volto a consentire, con un intervento e una presenza massiccia delle Forze dell'ordine, al Comune di Milano di completare il risanamento dell'area di Porto di mare, che - ricordo - era di 34 ettari che sono stati risanati. Restava, appunto, il boschetto, dove erano concentrate due piazze di spaccio che sono state, come sa il Presidente, Presidente, la piazza di spaccio per tutta la Lombardia. Prendiamo atto con soddisfazione che la nostra insistenza è stata premiata, che l'insistenza del Comune di Milano è stata premiata, che oggi le Forze dell'ordine sono intervenute in maniera massiccia e che ci sono le condizioni per risanare anche l'ultimo pezzo

di Rogoredo - che tra l'altro, ricordo, è stazione anche di transito e di sosta dei treni dell'alta velocità - è stato finalmente preso in carico. Si è aperta lo dico al Sottosegretario - la sede della Polfer e sono stati assegnati gli organici necessari. Tutto ciò va bene e approfitto di questo intervento per fare il passaggio successivo. Ora bisogna concludere il risanamento, ma diventa decisivo per la città evitare che, a questo punto, si spostino le piazze di spaccio e se ne creino altre nei quartieri limitrofi. quindi, che l'intervento a presidio di quei quartieri da parte delle forze dell'ordine debba essere mantenuto, proprio per evitare che l'effetto di un risultato molto positivo,

così come si è posto sul tavolo della prefettura il problema del contrasto allo spaccio, vi è anche un problema di aiuto ai tossicodipendenti e quindi di coinvolgimento dei servizi. Penso che si Penso che si stia andando nella direzione giusta e non bisogna assolutamente abbassare la guardia, ma occorre evitare che un fatto positivo si trasformi in un fatto negativo per altre zone della città. Su questo, oltre al Comune, che sta già operando, occorre che le Forze dell'ordine non siano smobilitate.

che presentano un alto indice di criminalità; nel suo ambito, infatti, sono presenti diversi immobili fatiscenti e in stato di abbandono, occupati anche da cittadini stranieri, alcuni dei quali risultano coinvolti in attività delinquenziali, in particolare nello spaccio di sostanze stupefacenti, nella prostituzione e nella vendita di merce contraffatta. A tal proposito, si rappresenta che nel suddetto quartiere lo scorso anno le forze dell'ordine hanno deferito all'autorità giudiziaria per spaccio di droga 37 stranieri, quasi tutti di nazionalità gambiana, molti dei quali appena diciottenni, contestando, altresì, 34 illeciti amministrativi per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nell'ottica di incrementare maggiori condizioni di sicurezza nella città e di contrastare, in particolare, il fenomeno dello spaccio di droga, il prefetto di Catania, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Catania e del sindaco metropolitano, ha provveduto all'elaborazione di una strategia volta ad incrementare l'attività di vigilanza del territorio, soprattutto concentrata in quelle zone che presentano un più alto indice di criminalità. A tal fine, proprio dal quartiere di San Berillo, nella notte del 22 novembre 2018, hanno preso avvio servizi straordinari e coordinati di controllo del territorio, con l'impiego di circa 80 unità fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, con il supporto dei militari impegnati nell'operazione Strade sicure, della Polizia municipale e dei Vigili del fuoco. La suddetta iniziativa ha consentito di sottoporre a controllo 70 persone e 29 mezzi; di rilevare 29 violazioni del codice della strada, con conseguente applicazione dì diverse sanzioni di carattere accessorio, quali sequestri e fermi amministrativi; di deferire all'autorità giudiziaria otto persone per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; di eseguire due perquisizioni in flagranza di reato; di procedere a tre sequestri di sostanze stupefacenti; di disporre la chiusura di alcuni esercizi commerciali per mancanza delle prescritte autorizzazioni e di irrogare le relative multe. Con cadenza periodica sono programmate in altri quartieri a rischio di Catania operazioni analoghe per riaffermare la presenza dello Stato nel territorio. Si informa, inoltre, che nei giorni scorsi si è conclusa nel quartiere San Cristoforo un'importante operazione di polizia giudiziaria denominata Stella cadente che ha portato all'arresto di 37 persone, 3 delle quali minorenni all'epoca

Signor Presidente, gentile Sottosegretario, cari colleghi, sono soddisfatta dell'esito dell'interrogazione e di aver appreso gli interventi messi in atto nella nostra città,

L'attività, se così vogliamo definirla, di questi ragazzi è infatti presente non solo nel quartiere di cui parliamo, ma in vari quartieri a rischio della zona del catanese.

Lo spirito della riforma si può riassumere nella volontà del legislatore di mantenere l'ente attuatore delle politiche governative d'internazionalizzazione nell'ambito delle pubbliche determinandone così una forte riduzione dei costi, affidata ad una nuova formula organizzativa più agile e più efficiente. È importante evidenziare che lo stanziamento totale del 2018 assegnato all'ICE è stato pari a circa 140 milioni di euro, mentre la somma di 177 milioni di euro citata nell'interrogazione parlamentare, si riferisce ad un totale che comprende più voci. Nel 2017, l'attività dell'ICE ha registrato la partecipazione di ben più di 19.000 aziende ad eventi promozionali organizzati per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. In questo contesto, sulla base di esigenze particolari dettate dalla situazione congiunturale, è emersa la necessità di aggiungere al fondo annuale per l'attività ordinaria dell'Agenzia ulteriori dotazioni finanziarie, disposte con apposite leggi volte a determinarne l'entità e le finalità specifiche. Per quanto riguarda il quadro delle risorse per il 2019, in particolare, rappresento che le risorse destinate al Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia sono passate da 130 a 140 milioni di euro. Sono sostanzialmente confermate le disponibilità di fondi per il Piano promozionale ordinario, per il Piano *made in Italy* e per il Piano *export* Sud. Nel complesso, quindi, nonostante i ben noti vincoli finanziari che hanno caratterizzato la costruzione della legge di bilancio per di cui siamo tutti al corrente, si é riusciti ad integrare già il più importante volano di risorse promozionali a sostegno dell'*export* per dare maggiore visibilità ai nostri prodotti nei mercati internazionali e favorire quindi il sistema Italia. Per quanto concerne invece le linee promozionali prioritarie per il 2019, la ripartizione delle risorse tra le diverse *macro*-iniziative è caratterizzata da alcune novità. luogo, un incremento delle risorse a sostegno del maggior utilizzo e della miglior visibilità delle imprese italiane su piattaforme e *marketplace* dell'*e-commerce* internazionale. il lancio del progetto innovativo High street Italia, che prevede l'allestimento di *show room* permanenti di sistema nelle principali capitali mondiali - il progetto pilota, che stiamo portando avanti, é in fase di avvio a Seoul, Shanghai e Osaka in cui concentrare e dare visibilità ai prodotti di qualità caratteristici del *made in Italy* di grandi *brand*, accanto a produzioni di piccole e medie imprese, uniti da uno *storytelling* comune, che esalti le caratteristiche di unicità storica, culturale e di gusto dello stile italiano. Il *budget* per questo tipo di iniziative di comunicazione è salito salito dai 16 milioni di euro dell'anno scorso ai 23 milioni di euro del 2019. In terzo luogo, una particolare attenzione al sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese *startup* e innovative, attraverso un progetto che, sul modello di quanto già realizzato con la misura dei *voucher* TEM (Temporary export manager), le sostenga nell'accedere ai servizi di importanti incubatori e acceleratori d'impresa all'estero. Per quanto riguarda il quadro delle missioni per il 2019, in attuazione e in programmazione, esse sono concordate e in linea con quanto deciso dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione e comprendono: missioni di sistema negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, Australia e Messico; missioni di *followup* in India, Vietnam, Brasile ed

Dunque, la differenziazione tra l'attività impostata a medio termine e la programmazione straordinaria permetterebbe al decisore pubblico di verificare tempestivamente se le politiche straordinarie di breve periodo hanno raggiunto l'obiettivo prefissato, rimodulandole Le direttive ministeriali espresse annualmente dalla cabina di regia interministeriale ed impartite all'Agenzia distinguono chiaramente, infatti, gli obiettivi di lungo periodo dell'azione in favore dell'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale da quelli di breve periodo, in genere a matrice settoriale o o geografica. La differenziazione dei fondi risponderebbe, quindi, anche all'esigenza di poter bilanciare la riprogrammazione delle iniziative. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, nello svolgimento della sua funzione di vigilanza, monitorerà costantemente l'andamento gestionale dell'ente, per conoscerne le effettive esigenze. La stessa riorganizzazione interna operata recentemente è infatti finalizzata al progressivo recupero di margini di efficienza dell'ente stesso e della sua attività.

sottosegretario Geraci. Ciò che ha detto va a rafforzare ancor di più la realtà e il lavoro che il Ministero dello sviluppo economico sta facendo in questi mesi nell'approcciarsi verso i mercati esteri. Lo sviluppo del *made in Italy* passa inesorabilmente attraverso l'attenta e puntuale valutazione dei singoli mercati esteri, ognuno con la sua specificità. L'*export* italiano negli ultimi anni ha fatto da traino per la nostra economia, gravemente colpita dalla crisi, contribuendo al mantenimento di interi settori produttivi. Io stesso, avendo una lunga esperienza nel settore ceramico, posso confermare come la crescita delle vendite al di fuori del nostro Paese sia stata fondamentale per la sopravvivenza di decine di aziende italiane. quindi, svolge questa importantissima funzione di raccordo, fornendo alle imprese italiane il *know how* di una grande agenzia nell'apertura di un canale extraeuropeo. L'Istituto ha contribuito negli anni all'internazionalizzazione di centinaia di aziende italiane con attività quali formazione, assistenza alle imprese, attrazione degli investimenti, comunicazione strategica, potenziamento delle filiere nazionali, organizzazione e intermediazione per fiere internazionali. Inoltre, nel grande mercato globale tutte le maggiori economie dispongono di agenzie specializzate per l'internazionalizzazione. Solo per citare alcuni Paesi, Francia, Brasile, Australia, Cina, Spagna, Germania, Giappone e Regno Unito hanno tutti agenzie che ottengono più del doppio dei finanziamenti del nostro Istituto per il commercio estero. Gli ultimi anni e le ultime legislature hanno purtroppo visto una trasformazione dell'ICE tutt'altro che positiva. L'ex ministro Calenda, con il suo piano straordinario per il *made in Italy,* ha spostato il finanziamento ordinario dell'ICE trasformandolo, appunto, in forma prevalentemente straordinaria, rifinanziata anno dopo anno. Proprio per tornare alla normalità nella pianificazione pluriennale delle attività dell'istituto è necessario tornare a finanziamenti ordinari sufficienti al funzionamento della sua struttura. Il ministro Di Maio ha dato un forte impulso in tal senso, innanzitutto con un grande impegno personale in missioni extraeuropee per favorire la crescita di *partnership* commerciali. Il mercato internazionale è duro e competitivo. Non dobbiamo affrontare questa sfida con paura, ma investendo e incentivando sempre di più le nostre imprese ad aprirsi a mercati nuovi al di fuori dei confini nazionali. La creazione di posti di lavoro passa anche da queste cose. Tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare, ma siamo sulla strada giusta.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la pubblica amministrazione.

trasporto pubblico locale e regionale

milioni di nostri concittadini "invisibili", che danno vita a un fenomeno che potremmo chiamare pendolarismo italiano perché riguarda la metà della nostra popolazione nazionale, nazionale, si imbattono, hanno a che fare e subiscono il nostro sistema di trasporto ferroviario locale, che versa ormai da tempo in condizioni estremamente critiche.

i ritardi, la mancanza di collegamenti diretti, le infiltrazioni, la presenza di insetti e topi, la scarsa illuminazione, i servizi igienici inagibili, i sedili sporchi, ambienti vetusti e la mancanza di riscaldamento e di sicurezza. Queste e tante altre sono le criticità che i viaggiatori si trovano a dover affrontare quotidianamente. A fronte dei numerosi annunci trionfalistici provenienti da esponenti dell'attuale maggioranza, manca un vero e proprio piano pluriennale efficiente di investimenti da realizzare a sostegno della mobilità.

Signor Ministro, una cosa non esclude l'altra. Noi siamo per le grandi opere. Voi potete anche essere contro, ma questo non esclude la riqualificazione della nostra rete ferroviaria regionale e locale, la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e prevenzione. A prescindere da come la chiamiamo - il TAV o la TAV - non dobbiamo far diventare quest'opera un alibi, un'arma di distrazione di massa. A farne le spese sono, come sempre, i nostri pendolari.

il senatore Ruspandini e gli altri interroganti. La prima cosa che dico è che non siamo contro le grandi opere. Siamo contro le grandi opere inutili e siamo totalmente, profondamente e ferocemente a favore delle grandi operi utili. Questo Governo ha impostato una linea di politica economica incentrata sul rilancio degli investimenti pubblici, al fine di stimolare l'economia del Paese e avviare una stagione di maggiore crescita economica e sociale. In particolare, oggi, il potenziamento del trasporto pubblico locale è uno degli obiettivi principali dell'azione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il programma di investimento sul trasporto pubblico locale relativo al periodo 2014-2033 è finanziato da fondi statali per oltre 13 miliardi di euro, oltre a un cofinanziamento regionale di circa 1,5 miliardi. Tali risorse sono destinate al rinnovo del parco autobus, al rinnovo del materiale rotabile per le ferrovie urbane, alla messa in sicurezza delle reti ferroviarie isolate e al potenziamento del trasporto rapido di massa. In particolare, a quest'ultimo fine sono state assegnate risorse, a valere sul fondo istituito con la legge di stabilità 2016, pari a circa 2,4 miliardi, che andranno a finanziare la realizzazione di progetti già nei prossimi mesi. Per quanto riguarda gli investimenti sulla rete ferroviaria nazionale, con il nuovo contratto di programma con RFI, valido fino al 2021, abbiamo destinato 2 miliardi per interventi di messa in sicurezza; quasi 700 milioni per investimenti in tecnologie per l'efficientamento delle linee e degli impianti; circa 1,3 miliardi per la valorizzazione delle reti regionali; quasi 900 milioni per il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture dei nodi metropolitani; circa 700 milioni per nuovi collegamenti con gli aeroporti e con i porti. L'attenzione verso i pendolari passa anche per il rinnovo della flotta regionale di Trenitalia, che ha già sostenuto 2 miliardi di investimenti per l'acquisto di 285 nuovi treni. Entro il 2024 saranno stanziati oltre 5 miliardi di euro per l'acquisto di nuovi treni. Con il prossimo aggiornamento al contratto di programma ulteriori risorse per circa 6 miliardi di euro saranno destinate agli investimenti ferroviari, la cui ripartizione terrà certamente conto delle esigenze dei territori e della necessità di ammodernare le tecnologie e innalzare i livelli di sicurezza. A titolo personale aggiungo che, una volta nominato il nuovo consiglio la prima cosa che dirò al nuovo amministratore delegato sarà di seguire il pendolarismo, i pendolari e l'efficientamento dei servizi a favore di chi quotidianamente, alzandosi la mattina presto e magari tornando la sera tardi, prende i mezzi di trasporto pubblico locale.

Presidente, ho ascoltato il Ministro con attenzione sia in Commissione che al *question time* alla Camera. Purtroppo, essendo pendolare, devo dire che la situazione non migliora. Mi auguro che ai buoni propositi facciano

il mio intervento tratta della messa in sicurezza di un movimento franoso che incombe sull'autostrada A5 presso il Comune di Quincinetto, al confine tra le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dove una frana di circa mezzo milione di metri cubi di roccia e detriti ha ripreso a muoversi negli ultimi mesi con una certa intensità, costituendo un serio pericolo per l'autostrada A5 Torino-Aosta con potenziali ricadute sull'abitato.

le misurazioni dei movimenti sono state rilevate anche attraverso un sistema di monitoraggio in tempo reale messo in atto a partire dal mese di ottobre 2018 dallo stesso Comune; risulta che il sindaco di Quincinetto, preso atto della situazione, ha chiesto, già da dicembre 2018, alla SAV, società incaricata della gestione del tratto autostradale, di controllare autonomamente i cambiamenti e gli spostamenti della frana, provvedendo alla segnalazione del pericolo ai viaggiatori e alla predisposizione di un piano d'intervento in caso di necessità, che prevede anche la chiusura del tratto autostradale che corre parallelo alla montagna; dai monitoraggi eseguiti le rilevazioni non avrebbero ancora evidenziato anomalie tali da rendere necessaria la chiusura del tratto autostradale; tuttavia, in caso di necessità, si dovrà valutare anche la chiusura per i potenziali pericoli per gli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A5 nella parte interessata dal movimento franoso; Da circa due anni è attesa la corresponsione di 4 milioni di euro da parte del Ministero competente per garantire la sicurezza dell'area. Il progetto è già stato approvato come intervento urgente nelle varie sedi. Si tratta di una grande opera per la messa in sicurezza di tutta l'area attraverso un sistema di terrazzamenti antifrana

Al fine di esaminare gli elementi acquisiti con il monitoraggio e l'individuazione di eventuali ulteriori iniziative finalizzate al contenimento del rischio, il Ministero dell'interno ha comunicato che nei prossimi giorni si terrà un tavolo tecnico con la partecipazione della prefettura di Torino, della Regione Piemonte, del Comune di Quincinetto e della concessionaria SAV. Quest'ultima ha già predisposto materiali e mezzi per la chiusura della tratta autostradale in caso di anomalie riscontrate dai sistemi di monitoraggio, misure che potranno essere eventualmente integrate dal predetto tavolo tecnico. Inoltre, la stessa società ha elaborato un progetto, oggi a livello di definitivo, che prevede un rilevato paramassi a protezione dell'asse autostradale; il progetto integra la sistemazione idraulica di un ramo della Dora e risolve anche alcuni problemi della viabilità secondaria nei tratti interferenti con l'autostrada. Infine, il Ministero dell'ambiente informa che sul sistema Rendis la Regione Piemonte ha già caricato l'intervento di difesa idrogeologica del versante in sponda destra del fiume Dora Baltea in località Chiappetti, per un importo richiesto pari a quattro milioni di euro. Per procedere all'erogazione dell'anticipo pari al 10 per cento, a luglio 2018 l'intervento è stato inserito nella banca dati unitaria (BDU) del MEF, e le risorse saranno a breve erogate. Concludo evidenziando che - sulla base di una preliminare relazione già predisposta dal Centro della Protezione civile - il sistema integrato di monitoraggio, i dispositivi di protezione fisica e le procedure di emergenza di protezione civile costituiscono un ottimale sistema armonizzato di prevenzione e intervento in caso di rischio. PRESIDENTE. *(L-SP-PSd'Az)*. Ringrazio il ministro Toninelli per la risposta, che dimostra la sensibilità di questo Governo per la messa in sicurezza dei nostri territori e delle nostre reti viarie. Non dimentichiamo che il tratto di collegamento autostradale di cui stiamo parlando è un'importante arteria di collegamento veloce tra Torino e Aosta ed è un'arteria indispensabile per il settore turistico in qualsiasi stagione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, porto oggi all'attenzione dell'Assemblea una questione importante, relativa ad opere e cantieri, e quindi al lavoro. Lo scorso 15 novembre, in Conferenza unificata, in Conferenza unificata, è stata approvata un'intesa del cosiddetto piano di rientro strade, in cui si intende riclassificare come strade di interesse nazionale, e dunque a gestione ANAS, 2.713 chilometri di tratte regionali e provinciali, di cui,

ma che è ferma a Carceri ormai da più di trent'anni. Mancano sette chilometri da Carceri allo svincolo della A31; 10 chilometri per arrivare a Montagnana; serve circa 220.000 abitanti. Si tratta di un piccolo intervento, Ministro, Ministro, piccolo, piccolissimo. Non parliamo di grandi opere, ma di opere essenziali per la vita e lo sviluppo di quei territori; per lo sviluppo delle nostre aziende ma anche per ognuno di noi, per le famiglie, per chi ci abita, per avere un futuro, per i nostri giovani. Sono stati portavoce di questa battaglia sindaci, amministratori locali, persone di tutte le categorie economiche, associazioni, comitati di cittadini di tutti i colori, non di appartenenze partitiche ma di tutti i colori di quel territorio. Il territorio dove incide la strada regionale 10 è particolarmente colpito da una grave crisi economica e occupazionale ed è fondamentale completare quest'opera per attrarre investimenti, per far arrivare nuove aziende e far sì che quelle attuali non chiudano ma possano avere un futuro. riqualificare le zone industriali e artigianali della Bassa Padovana, che è stata dichiarata, purtroppo, area di crisi non complessa (distretto, ad esempio, del mobile di Casale di Scodosia, dell'agroalimentare del Montagnanese ), è fondamentale, direi essenziale,

chiedendo proprio, in modo particolare, la realizzazione del primo stralcio funzionale della SR10. La Regione Veneto, attraverso il presidente Zaia, ha già messo le risorse

no alla strada regionale 10, un minuscolo intervento, un «microbo», se così possiamo definirlo, però fondamentale per lo sviluppo di quel territorio.

alla luce delle forti asimmetrie territoriali conseguenti alla riclassificazione derivante dalla riforma Bassanini, nonché dei fallimentari effetti della riforma Delrio sulle Province. *(Commenti dal Gruppo PD).* Il decreto del Presidente del Consiglio del 21 Luglio 2017, in applicazione dell'articolo 1, della legge di stabilità del 2016, ha stanziato nel Fondo infrastrutture 440 milioni destinati a interventi di riclassificazione della rete stradale. Successivamente, nel 2018 il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato per oltre 640 milioni di euro. Ad oggi, quindi, per gli investimenti sui tratti stradali trasferiti dalle Regioni ad ANAS sono stanziate risorse pari ad oltre un miliardo di euro. Il decreto con cui la Regione Veneto ha trasferito circa 700 chilometri di strade ad risulta attualmente in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; quindi, abbiamo terminato l'*iter*. Nel prosieguo dell'*iter* in corso, il Ministero porrà la massima attenzione per un'opera strategicamente importante

Signor Ministro, ad oggi 13 Regioni a statuto ordinario su 15 hanno avviato la procedura per il riconoscimento di maggiore autonomia rispetto allo Stato centrale. Paradossalmente, però, sulla nutrita schiera di richieste grava l'assenza di quella che dovrebbe essere la bussola di questi processi: mi riferisco alla definizione di criteri uniformi che presiedano alla singola valutazione e di procedure idonee a conseguire un accordo complessivo con tutte le Regioni a statuto ordinario sugli strumenti di perequazione delle risorse. Ma non basta. A corredo di queste due marchiane assenze, ci sono ulteriori criticità. La prima è quella che investe il ruolo e la funzione del Parlamento, che non può continuare ad essere il convitato di pietra delle intese. La seconda invece riguarda il troppo fumoso precipitato degli esiti di questi differenti *iter* di differenziazione. Riguardo al primo punto, signora Ministro, mi limito a ricordare la *ratio* del comma 3 dell'articolo 116, dove le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite con legge dello Stato. Capisco che volete ormai farci abituare al progressivo svuotamento della funzione legislativa in capo al Parlamento; lo abbiamo visto con la legge di stabilità ce lo avete riproposto con il decreto milleproroghe e "mille rivoli". Ma le leggi dello Stato devono quantomeno essere lette, eventualmente emendate, e poi, solo poi, approvate dalle due Camere. Nella giornata di ieri è arrivato l'appello di 30 costituzionalisti, inviato al presidente Mattarella e ai Presidenti di Camera e Senato, nel quale viene ribadita questa forte preoccupazione per le modalità di attuazione finora seguite e per il rischio concreto di una marginalizzazione del Parlamento, che è - lo ricordo - l'unico luogo di tutela degli interessi nazionali. Oltre a chiederle, signor Ministro, quali sono gli intendimenti dell'Esecutivo su tale ambito, intendo far presente anche l'esigenza di una pre-intesa. Non è possibile infatti che ci sia una modifica costituzionale fatta senza sentire le altre Regioni, perché anche le altre Regioni sono parte di un accordo necessario. Sono messe in discussione infatti le istituzioni dell'uguaglianza, *in primis* in tema di salute, istruzione e protezione sociale, che servono a realizzare il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione e che necessitano di una decisione corale e di una partecipazione vera alla decisione. Anche qui, signor Ministro, in che modo e quando questo Governo si produrrà nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni? È una scelta che va fatta a monte non a valle. Non possiamo infatti legare questi diritti al reddito dei residenti; non si può legare la cittadinanza e la possibilità di esercitare i propri diritti al luogo di residenza. Mi sia permesso infine, signor Presidente, un brevissimo inciso. Personalmente, insieme a tante migliaia di cittadini, ho sottoscritto la petizione del professore Viesti, che, ben argomentando nei fatti, sintetizza questi maggiori poteri, in special modo al Veneto e alla Lombardia, come la secessione dei ricchi. PRESIDENTE. Ed è una secessione che avviene solo in apparenza con i guanti di velluto, perché sostanzialmente questo Governo sta tentando di mettere la parola fine, la pietra tombale su quella che è già la nostra Italia

continuo a ricordare che, nell'ambito dell'autonomia differenziata, stiamo parlando dell'attuazione di una previsione costituzionale. Così come indicato dalla norma, si prevede che le competenze siano attribuite con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Il ruolo che quindi la Costituzione attribuisce al Governo nell'*iter* delineato nella previsione costituzionale è semplicemente quello di trovare l'intesa rispetto alle richieste avanzate dalla Regione. In questa fase, com'è noto, l'Esecutivo sta completando un'intensa e complessa attività istruttoria e di negoziazione, che è propedeutica alla redazione di un testo o, meglio, di uno schema di testo condiviso con le Regioni. Il Governo è assolutamente disponibile ad aprire un confronto con il Parlamento in merito al contenuto di questo progetto, nelle forme che verranno definite ovviamente nel rispetto delle prerogative del Parlamento. Il Governo è ben consapevole della centralità delle Camere nell'ambito di un processo di trasferimento di competenze legislative che assume un rilievo costituzionale e che vede il Parlamento doverosamente coinvolto. Per quanto riguarda le altre Regioni richiedenti l'autonomia differenziata, abbiamo definito un testo relativo alle richieste della Regione Piemonte, che mi appresto ad inviare a breve a tutti i Ministeri competenti. Oggi, tra l'altro, ho incontrato il presidente De Luca per avviare l'istruttoria sulle richieste della Regione Campania. Sul quesito di trattare in modo congiunto le richieste delle Regioni, devo osservare che tale ipotesi non trova riscontro di fattibilità. Le richieste di autonomia sono arrivate in momenti diversi: le prime, quelle di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, sono partite addirittura nella precedente legislatura e hanno portato ad un pre-accordo firmato dal Governo Gentiloni Silveri, per cui è come se ci fossero delle velocità diverse. Successivamente sono pervenute le richieste di Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche e, nel mese di gennaio, quella della Campania. Le domande di autonomia sono eterogenee per materie e competenze. È comunque compito del Governo garantire un impianto generale identico per tutte le richieste di autonomia.

Per quanto riguarda la richiesta di definire preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni, ricordo che le bozze di intesa richiamano al loro interno, sia i fabbisogni *standard*, sia i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assolutamente realizzati. La definizione

per il nostro Paese questa consapevolezza risieda nelle argomentazioni che oggi state portando avanti, specialmente nel momento in cui manca la definizione di tutta una serie di elementi, come lei ha dimostrato in questo momento, dai fabbisogni *standard,* alla definizione dei LEP, ad una definizione anche in rapporto alla capacità fiscale dei territori. Tutti questi elementi mancano, per cui siamo davanti ad un rapporto bilaterale tra il Governo e le Regioni per definire delle intese che non sappiamo in quale tipo di equilibrio potranno stare rispetto al bilancio dello Stato e alla

che non porterà da nessuna parte nella definizione dell'autonomia e delle richieste di regionalismo differenziato che sono state fatte.

nelle attuali tre bozze di intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, datate 25 febbraio 2019 e pubblicate sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, è prevista l'applicazione automatica, dopo tre anni, della spesa media nazionale. Le formule per il trasferimento di risorse al Veneto, alla Lombardia e all'Emilia-Romagna prevedono che, per ciascuna voce, l'ammontare delle risorse assegnate non possa essere inferiore al valore medio nazionale *pro capite*.

una concentrazione della spesa che aumenta i già presenti squilibri economici in favore delle Regioni più ricche. Sul sito del Dicastero per gli affari regionali è pubblicata una tabella con la spesa *pro capite* per l'istruzione universitaria in alcune Regioni, dove al vertice viene indicata l'Emilia-Romagna, con 163 euro, e in coda la Puglia, con 93 euro. A dispetto delle dichiarazioni del Ministero in indirizzo in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle bozze di intesa Stato-Regioni del 25 febbraio scorso non c'è alcun passaggio che leghi il trasferimento di funzione e risorse, né tanto meno il calcolo dei fabbisogni *standard*, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni pur Sul sito del Ministero è stata pubblicata una tabella con i confronti territoriali nella spesa statale, che vedono Lombardia e Veneto in coda alla classifica della spesa *pro capite.* La fonte è la Ragioneria generale dello Stato, che tuttavia visiona appena un quarto della spesa del settore pubblico, mentre la banca dati dei conti pubblici territoriali, che fa capo al MEF, non è stata considerata in alcun modo nonostante sia stata pensata proprio per verificare l'azione del sistema pubblico nelle Regioni. Considerato che i dati dei conti pubblici territoriali permettono di raffrontare in maniera affidabile la distribuzione della spesa nelle diverse Regioni e dimostrano come la spesa pubblica complessiva sia sensibilmente più elevata per le Regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Mezzogiorno, il rapporto 2018 sui conti pubblici territoriali riporta che la spesa *pro capite* nel settore pubblico nel suo insieme si attesta a 15.000 euro per le Regioni del Nord contro i 12.000 euro per quelle del Sud. Si chiede, pertanto, di sapere: se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di pubblicare una tabella di raffronto sulla spesa statale per le Regioni che prenda come riferimento i dati dei conti pubblici territoriali; se la pubblicazione nei confronti di spese relative alle università sia la premessa per una riduzione di risorse destinate agli atenei dell'Emilia-Romagna, in favore in particolare di quelli della Puglia; se non sia opportuno tralasciare l'aggancio automatico alla spesa media *pro capite*, portatore di ulteriori squilibri nel bilancio statale, in ragione di altre metodologie di calcolo che facciano riferimento a una pur tardiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni *standard*.

alla luce dei continui incontri con i vari Ministeri e di quanto risulterà anche dal confronto con il Parlamento. La scheda riportata sul sito fa riferimento alla spesa statale regionalizzata pubblicata dalla Ragioneria generale dello Stato ed è la spesa relativa ad alcune funzioni statali esercitate nelle Regioni. Poiché l'oggetto dell'autonomia differenziata è l'attribuzione alle Regioni di competenze legislative e amministrative dello Stato, il tema della quantificazione delle risorse finanziarie non può che essere strettamente collegato alla spesa attuale dello Stato per l'esercizio delle funzioni da trasferire.

l'onorevole senatore, pur avendo rilevanza sul tema della spesa nei territori, non hanno una relazione con le funzioni da attribuire alle Regioni in base all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tali dati riguardano il complesso della spesa pubblica nelle Regioni, comprendendo anche quella degli enti territoriali e delle aziende pubbliche, quindi non inerente al calcolo necessario per determinare le risorse derivanti dall'attribuzione di competenze statali. In realtà, quando queste competenze saranno definite, la quantificazione delle risorse necessarie sarà determinata rilevandole dai bilanci dei Ministeri coinvolti, individuando così le spese che attualmente gli stessi sostengono per lo svolgimento della funzione nel territorio regionale. Il valore, quindi, è un dato oggettivo certo e non avrà, né deve avere, alcun impatto complessivo sul bilancio dello Stato. Ricordo che l'intesa deve essere sottoscritta senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda il riferimento alla spesa universitaria, nella scheda pubblicata sul sito del Dipartimento è stata riportata tale voce solo a titolo esemplificativo. La bozza d'intesa non prevede in alcun modo un ipotetico trasferimento di risorse relative al fondo di finanziamento ordinario. Anche se non sarebbe necessario, ribadisco una cosa scontata: nelle bozze dell'intesa l'autonomia delle università non è assolutamente Per concludere, ricordo che nell'intesa definitiva, con l'individuazione precisa delle materie e delle competenze da trasferire, potremmo individuare la spesa storica, di concerto con il MEF. Per noi resta primaria la definizione dei fabbisogni *standard* unitamente ai livelli essenziali delle prestazioni, ai fini dell'efficientamento della spesa, ma in contestuale garanzia di un'erogazione omogenea di servizi su tutto il territorio nazionale.

da oggi: è un argomento ricorrente negli ultimi diciannove anni. Siamo certi che il procedimento verrà attuato nel rispetto dei valori portanti della coesione e della solidarietà, quindi secondo i principi richiamati dalla nostra Costituzione. *(Applausi

In sostanza, la combinazione tra quota 100, i pensionamenti ordinari, la legge di bilancio con il relativo, al netto della scuola e delle Forze dell'ordine, blocco delle assunzioni

che parlano sostanzialmente di un fabbisogno di 150.000 cattedre e di circa 24.000 posti ATA,

Se così fosse, la situazione critica in cui ci siamo trovati nell'anno scolastico attuale, nel prossimo anno esploderebbe in modo drammatico

tra Governo e Regioni sui *navigator*, perché gli *spot* vanno bene, ma se c'è un conflitto non capisco come riuscirete a gestire questa partita

unità, a cui si aggiungono le 150.000 presentate dagli aventi diritto a pensione secondo i requisiti della legge Fornero. Queste sono le stime, ma si tratta di dati che erano ampiamente previsti, che ritengo

adottata una serie di provvedimenti: mi riferisco alle disposizioni che consentono di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, in misura pari al 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente; all'utilizzazione di graduatorie vigenti e alla possibilità d'indire nuovi concorsi senza autorizzazione preventiva (questa è la cosiddetta SCIA per le assunzioni); ad assunzioni straordinarie, di cui pochi parlano, ma che credo siano importantissime, utilizzando risorse stanziate nell'ultima legge di bilancio (pari, nel triennio 2019-2021, a 893 milioni di euro, per la maggiore parte già distribuiti tra le varie amministrazioni). Aggiungo che durante l'esame del disegno di legge cosiddetto quota 100, sono stati presentati dal Governo e già approvati al Senato alcuni emendamenti che nel triennio nel triennio 2019-2021 consentiranno alle Regioni e agli enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per cinque anni e di conteggiare, ai fini della programmazione di quelle nuove, le cessazioni dal servizio che si verificheranno in corso d'anno; al Ministero della giustizia di assumere, secondo modalità semplificate, a partire da luglio, 1.300 unità; alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie dei nuovi concorsi espletati per assumere i vincitori ed eventualmente sostituirli, fermo restando l'ordine di merito. Possiamo quindi dire che gli effetti dei pensionamenti verranno compensati dai nuovi concorsi e dall'utilizzazione delle loro graduatorie. In particolare, visto che il tempo sta finendo, per quanto riguarda

le graduatorie contengono 33.000 unità. L'ultimo dato che le fornisco è che è intenzione del Governo presentare un emendamento che consentirà alle aziende e agli enti del servizio sanitario di conteggiare, ai fini delle nuove assunzioni, al pari di Regioni ed enti locali, anche le cessazioni dal servizio che si verificano in corso d'anno. Per quanto riguarda i *navigator*, c'è una confusione generale: non sono pubblica amministrazione, quindi non rientrano nella mia competenza, ma non c'è alcun conflitto.

Le assicuro che purtroppo non è così. In secondo luogo, le chiederei di approfondire un po' di più l'incrocio terribile tra le norme in relazione alle assunzioni in sanità,

consiglierei di mettere insieme tutte le norme: scoprirà che il combinato disposto mette in crisi il sistema. Non parliamo poi dei concorsi: davvero pensate che i concorsi in questi mesi risolveranno il problema drammatico in cui ci troviamo? Secondo me, signor Ministro, siete un po' troppo tranquilli. Dovete trovare degli strumenti straordinari, superare i vincoli, sburocratizzare il meccanismo delle assunzioni e aprire una nuova fase. In relazione ai *navigator*, so bene che non sono di sua competenza e le chiedo scusa; tuttavia, visto che rappresenta il Governo, l'unica cosa che non mi può dire è che non c'è un conflitto tra le Regioni e il Governo. una cosa sancita e definita con grande chiarezza. Le ribadisco dunque la preoccupazione e le chiedo di fare un approfondimento.

Signor Presidente, gentili senatrici e senatori, intervengo oggi in Aula per ricordare e chiedere, alla fine del mio intervento, un minuto di silenzio per Carmelo D'Addetta, un agente di polizia locale di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Sono qui presenti oggi, per assistere alla seduta, i suoi familiari, il sindaco di San Nicandro e alcuni rappresentanti della polizia locale. Nel giorno di Ferragosto dello scorso anno, Carmelo D'Addetta venne travolto da un'auto in corsa, mentre era impegnato nei rilievi di un tragico incidente stradale, avvenuto poco prima sulla strada statale 693, in cui avevano perso la vita due giovani ragazze e un ragazzo di Torremaggiore. Dopo mesi di ricovero in ospedale, Carmelo è venuto a mancare il 13 novembre. Sono venuta a conoscenza di questa tragica vicenda lo scorso gennaio, quando ho partecipato al convegno nazionale del Sindacato unitario dei lavoratori della polizia locale (SULPL). Al convegno nazionale del SULPL, alla presenza dei familiari, l'agente D'Addetta ha ricevuto un attestato e una medaglia d'oro alla memoria, per aver pagato con la vita la sua grande dedizione e l'attaccamento al lavoro. Purtroppo lo Stato spesso si dimentica di tali uomini e donne che svolgono un importante servizio a favore della comunità e della cittadinanza locale contro il crimine, nel contrasto a reati, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti e la prostituzione, e nella tutela dell'ordine pubblico. Spesso, essi si trovano ad affrontare situazioni critiche e di disagio, ad alto impatto emotivo senza nessun supporto anche psicologico. Nel caso di agenti di polizia locale, le morti per cause di servizio rimangono spesso anonime; esse meritano al contrario un segno di attenzione da parte delle istituzioni e, nel nostro caso, del Parlamento Il MoVimento 5 Stelle ha già presentato un disegno di legge a prima firma del collega, senatore Corbetta, per l'estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo. Tale estensione rappresenta un atto doveroso da parte dello Stato, proprio in nome dei principi fondamentali tutelati e riconosciuti dal nostro ordinamento, che non può tollerare *status* normativi diversi in relazione alle differenti modalità nelle quali il sacrificio della vittima si è consumato. Sarebbe un primo riconoscimento a chi offre e ha offerto, anche a costo della vita, tale alto servizio al Paese, con onore e dedizione. Gentile Presidente, colleghe e colleghi, in conclusione chiedo quindi a tutta l'Assemblea di offrire un segno tangibile di vicinanza a questi lutti,

il 9 marzo 1945 furono trucidati sette partigiani. Da allora c'è un ricordo continuo e costante, che si celebra con una particolare sensibilità, estesa a tutto il territorio. La storia di per sé è drammatica. Quest'anno a Pessano con Bornago il 17 marzo è stato organizzato - e non ci vediamo nulla di male - un evento sportivo da combattimento che vede come protagonista l'associazione Wolf of the ring (WTR) a sostegno della ONLUS Bran.Co. Sia l'associazione che la ONLUS in questione fanno riferimento all'organizzazione di estrema destra Lealtà Azione; Bran.Co è stata al centro di recenti polemiche perché sembra che nella propria attività di aiuti a famiglie in difficoltà abbia messo in atto azioni di vera e propria discriminazione nei confronti delle famiglie non italiane. L'ANPI di Pessano con Bornago si è accorta che questa manifestazione privata sportiva è patrocinata dalla Regione Lombardia. L'unica cosa che ANPI ha chiesto, senza voler fare eccessivo rumore, ma sottoponendo, secondo la formula più democratica, una sorta di ordine del giorno anche a tutti i Comuni limitrofi per trovare un sostegno, che la Regione Lombardia tolga il patrocinio. Si tratta di una manifestazione fatta in un luogo privato, oltretutto in un luogo che, forse, il buon senso e anche il buon gusto, visto poi il mese in questione, dovrebbe vedere

che la Regione, che, tutto sommato, è una Regione di tutti, anche dei cittadini che non si sentono da questa manifestazione rappresentati, possa scegliere in questo modo, così palese, di sostenere un evento

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, molti di voi avranno letto l'editoriale di Tomaso Montanari, pubblicato martedì 5 marzo su «il Fatto Quotidiano», dal titolo «L'indegna apologia del ladro di libri». Montanari, ottimo storico dell'arte e noto protagonista del dibattito culturale italiano, prende nettamente le distanze dall'ultimo saggio del professore Sergio Luzzatto, ordinario di Storia moderna presso l'Università di Torino, che per i Tipi di Einaudi ha appena pubblicato il saggio «Max Fox o le relazioni pericolose». Chi pensasse, giudicando dal titolo, ad un'avventura di Geronimo Stilton o di Harry Potter cadrebbe in un tragico errore. Ho detto tragico, invece dovrei dire tragicomico, perché la trama dello scritto di Luzzatto, un saggio appunto, non una novella, non è di fantasia, ma si ispira ad un fatto gravissimo, una storia italiana che rasenta il ridicolo nella sua drammaticità e che, se non fosse cosa giudicata, apparirebbe incredibile: la biblioteca dei Girolamini di Napoli depredata dal suo direttore, Marino Massimo De Caro. Al sequestro della biblioteca e all'arresto del De Caro, presunto campione del commercio illecito di libri su scala internazionale, arrivato nel 2011 alla direzione di uno dei più importanti presidi culturali italiani per una congiunzione astrale favorevole, evidentemente (ma forse non è superfluo ricordare che, questa volpe, messa a guardia del pollaio, come scrive Montanari, Montanari, era il braccio destro di Marcello Dell'Utri, uomo di Publitalia, proprio come l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali, Giancarlo Galan). Seguì la condanna a sette anni per peculato, mentre pende tuttora il giudizio per associazione a delinquere, devastazione e saccheggio. Se in Italia la devastazione e il saccheggio del patrimonio culturale pubblico, appunto, non sono stati ancora legalizzati, come si spera che la sentenza possa in futuro ribadire, nessun dubbio è ammissibile sulla liceità, ma neppure sulla inopportunità, di dare dignità letteraria e, più o meno esplicitamente, assolvere, com'è palese fin dal titolo sussiegoso del saggio di Luzzatto, il protagonista di imprese truffaldine particolarmente odiose, perché tese a depauperare i nostri beni culturali. Si è molto discusso, colleghi, del valore diseducativo di certe produzioni cinematografiche e, più di recente, di certe *fiction* sulla criminalità organizzata, fortunatissime quanto ai numeri e al gradimento del pubblico, ma accusate di attenuare la riprovazione sociale nei confronti di quelle devianze e, peggio, di trasformare i protagonisti in eroi, fino a suscitare emulazione. Ebbene, non è meno grave che il professor Luzzatto, neo ufficio stampa del novello Lupin, si faccia complice di un reato odioso come quello commesso a danno dell'eredità culturale del Paese, materializzata nel patrimonio librario. L'avrà ispirato il fascino del crimine o, piuttosto, un furbesco ammiccamento al lettore che, notoriamente, nell'eterna lotta tra guardie e ladri, sotto sotto parteggia per i secondi? Stupisce una scelta simile da parte di un docente universitario. Stupisce, ancor di più, che un editore di altissimo profilo come Einaudi si sia prestato, per mero profitto, ad un gioco così sporco. Bene ha fatto Tomaso Montanari, già autore della denuncia pubblica che innescò l'indagine, a bollare l'iniziativa editoriale come «L'indegna apologia del ladro di libri».